Comunico che in data 5 dicembre 2023 è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il seguente disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18

Grazie recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei

Ci deve dire qualcosa sulle premesse, però.

favorevole con riformulazione di ciascun impegno. Quindi tutti gli impegni devono essere riformulati aggiungendo le parole: «a valutare l'opportunità di» (...) «compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica».

esprimo parere favorevole con riformulazione dell'impegno in «a valutare l'opportunità di» (...) «compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica». Solo questa modifica, Presidente.

del secondo impegno: «ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, per affrontare il nodo dell'abusivismo edilizio».

riformulazione del secondo impegno: «ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, per affrontare il nodo dell'abusivismo edilizio».

favorevole con riformulazione dell'impegno in «a valutare l'opportunità di» (...) «compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica».

di tutti quei cittadini al cui controllo dell'immobile non viene certificata l'idoneità alla sismicità. In tal caso i cittadini andrebbero incontro

6. Colleghi, da questo momento siamo nei tempi giusti per poter iniziare le operazioni di esame e di voto degli emendamenti. Essendone

si tratta di un modo di procedere poco utile ad affrontare le cose. Il provvedimento ha degli aspetti positivi e anche degli aspetti che ovviamente ci preoccupano. Ho chiesto la parola sull'articolo 6 perché è uno dei punti di preoccupazione rispetto al decreto-legge in esame, la funzione di avviare una capacità di prevenzione (un termine un po' eccessivo) o di intervento, al fine di evitare che una situazione sempre più preoccupante possa degenerare e lo fa attraverso la scelta di lavoro delle persone, necessità di informazione e di mettere al riparo, di avere la strutturazione.

Io credo che ci sia uno iato tra il senso del decreto-legge (la presa in carico di una situazione difficile) e le risposte che poi si danno sul terreno del lavoro e dell'occupazione, che non sono mai all'altezza degli impegni che vengono richiesti. Tutto ciò sapendo che parliamo di un'area,

perché non ci sono. Bisognerebbe quindi, come sempre, se si vuole davvero fare prevenzione, investire anche nelle capacità professionali, nel personale e nell'occupazione, sostenendo quei Comuni che sono in difficoltà. L'emendamento 6.1 è ovviamente parziale rispetto all'insieme delle cose che ho detto, ma sarebbe un segnale importante per dimostrare che il senso di questo decreto-legge viene anche sostenuto dalle scelte occupazionali che si fanno.

il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge, su proposta del presidente Giorgia Meloni e del ministro Nello Musumeci, mirato a prevenire il rischio sismico causato dal fenomeno del bradisismo nell'area dei Campi Flegrei, una zona vulcanica molto estesa. Il decreto-legge permette l'adozione di un piano straordinario per valutare la vulnerabilità delle zone edificate colpite da questo fenomeno. L'onere finanziario complessivo quantificato per arginare queste minacce è di 52,2 milioni di euro, che saranno coperti integralmente dallo Stato. Nella zona dei Campi Flegrei l'attività sismica causata dal bradisismo non accenna a diminuire. Scosse sismiche si verificano con frequenza crescente, tra cui una di magnitudo 2.6 alle ore 10,46 del 4 ottobre, seguita da un'altra di magnitudo 1.7. Questa situazione sta causando crescente preoccupazione tra i residenti. residenti. I Comuni della zona, nonostante abbiano affrontato il bradisismo per più di un secolo, non dispongono però ancora di piani di evacuazione specifici per gestire questa minaccia. decreto-legge Campi Flegrei contiene le disposizioni per l'adozione di un piano di emergenza straordinario che comprende quattro attività principali: uno studio di microzonazione sismica, l'analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia privata, l'analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia pubblica, con misure di mitigazione, e un programma di monitoraggio sismico e delle strutture. Il Dipartimento della protezione civile delineerà urgentemente l'area di intervento basata sui dati di sollevamento bradisismico e sismicità. Per implementare il piano in modo rapido il Dipartimento disporrà di un supporto speciale. Inoltre, un piano di comunicazione alla popolazione, in coordinamento con la Regione Campania e il Dipartimento della protezione civile, mira a sensibilizzare la popolazione sui rischi sismici, con un'attenzione particolare alle persone con disabilità. Entro sessanta giorni verrà elaborato un piano di emergenza per l'area interessata dal bradisismo, basato sui dati dei centri di competenza e contenente procedure per situazioni di emergenza. Saranno attuate inoltre misure per verificare l'integrità delle infrastrutture di trasporto e altri servizi essenziali. Sotto la coordinazione della Regione Campania, verrà potenziata la risposta operativa territoriale di protezione civile. La Città metropolitana di Napoli coordina sforzi per reclutare personale temporaneo, acquisire i materiali necessari e allestire strutture temporanee per l'accoglienza della popolazione. Il piano deve considerare la decisione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di mantenere il livello di allerta giallo per il rischio vulcanico. Inoltre, per quanto riguarda la sismicità legata al bradisismo, la Commissione ha notato un aumento nella frequenza e nell'intensità degli sciami sismici, suggerendo la possibilità di eventi sismici futuri simili. Gli scienziati raccomandano una serie di misure per affrontare il rischio sismico nei Campi Flegrei. Queste misure includono la riduzione significativa della popolazione residente nella zona rossa, che conta circa 600.000 persone; l'implementazione di uno schema di evacuazione progressiva, iniziando da una piccola area considerata ad alto rischio; l'evacuazione temporanea degli edifici situati entro un chilometro e mezzo dall'area della Solfatara Agnano, dove si verificano i terremoti più intensi, per valutare la loro abitabilità e resistenza a scosse sismiche significative. Gli esperti sottolineano l'importanza di sviluppare un piano di evacuazione specifico per il rischio flegreo, che è complesso e include il rischio di eruzione vulcanica. Siamo vicini ai cittadini dei Campi Flegrei colpiti da questa terribile minaccia. Al legittimo sgomento delle persone costrette ad abbandonare le loro case in piena notte a causa dell'aumentare significativo dell'attività sismica dovuto al fenomeno del bradisismo, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha risposto prontamente con il decreto-legge che stanzia 52,2 milioni di euro per permettere la messa in sicurezza dei territori interessati dal rischio eruzione. Riteniamo prioritaria la coordinazione a più livelli istituzionali di tutti gli enti interessati per coordinare un piano di emergenza che possa efficacemente salvare i cittadini da un fenomeno sismico o eruttivo purtroppo non del tutto prevedibile. La sfida è proprio farsi trovare pronti a questa terribile eventualità. Di fronte alla messa in sicurezza dei cittadini e delle infrastrutture, nessuna polemica politica deve rallentare o disturbare la collaborazione tra Protezione civile, Regione Campania, Città metropolitana e comunità scientifica. Una volta certi della sicurezza dei cittadini, si potrà indagare sui motivi per cui fino ad ora non sono stati attuati provvedimenti per far fronte a un fenomeno ciclico e secolare come quello del bradisismo che interessa la zona vulcanica dei Campi Flegrei.

che i Campi Flegrei siano un territorio soggetto da sempre a fenomeni sismici è cosa nota. Ci sono state alcune recrudescenze negli ultimi tempi, per cui è ovvio che si debba intervenire

al Parlamento come provvedimento preventivo. Abbiamo parlato sempre di fare prevenzione: adesso la si fa e, quindi, va bene ma va davvero bene? Ora, i colleghi toscani mi perdoneranno, ma

perché l'è tutto sbagliato, l'è tutto da rifare? Come si fa a pensare che si possa davvero realizzare in novanta giorni un piano di misure urgenti di prevenzione dal rischio sismico in cui sono coinvolti undici enti diversi, più il Commissario straordinario di cui all'articolo 5, comma 2-*bis*, dei quali uno è la Regione Campania, che evidentemente ha più uffici coinvolti, e gli altri sono i Comuni della zona, che sono certamente più di uno? Voi pensate che a mettere intorno a un tavolo in

È chiaro che non possiamo militarizzare tutto l'apparato pubblico statale italiano, ma qualcosa di meglio si può fare, come dimostrano anche altri apparati pubblici del nostro Paese: cito quelli che conosco, le autonomie, cui apparati c'è una chiara distinzione tra chi fa cosa. Pertanto, un piano speditivo si farebbe in cinque giorni, perché non c'è bisogno di mettere d'accordo tutta una serie di soggetti che hanno competenze complesse che - come detto - si sovrappongono tra loro. questo provvedimento si utilizzano cinque volte le parole «celere» e «speditivo»: ha senso continuare a ripetersi di dover essere veloci? Ha senso, sì, perché in questo modo si mettono le mani avanti. Tenete conto che qui tutte le attività operative vengono demandate all'ente locale; la Regione e i Comuni si devono occupare del monitoraggio e della determinazione dei fabbisogni, e cioè gli apparati dello Stato coordinano, indirizzano e controllano. È abbastanza comodo fare questo, senza l'assillo di dover operare, perché chi opera sono gli altri. Anche in questo provvedimento, quindi, assistiamo al *cliché* tipico dello Stato italiano, tale per cui lo Stato non si assume responsabilità operative, che sono quelle che chiedono il tempo, e lascia con la faccia nel vento gli enti locali.

Quali strumenti e quali agevolazioni fiscali si metteranno a disposizione di questi cittadini, per mettere in sicurezza le loro case? E poi, quanto alle vie di fuga, su quell'area insistono e abitano 550.000 persone e, quindi, si deve porre il tema delle infrastrutture: se devono allontanarsi velocemente, dovranno avere le strade per poterlo fare e anche di dimensioni adeguate. Lo sono? C'è qualcuno che si preoccupa degli investimenti conseguenti? Insomma, si tratta di un provvedimento farraginoso, centralizzante e privo totalmente di agilità delle procedure. Come ho detto all'inizio, plaudo al fatto che ci sia un provvedimento preventivo, ma è un provvedimento che così non può funzionare. Dunque il mio auspicio è che, su questa base, si possano apportare in futuro migliorie per rendere sempre più agile ed efficace la catena di comando e per far sì che il piano di comunicazione, che ricopre un'importanza assoluta, risponda alle necessità. Qui siamo un po' in una situazione campata per aria e, come al solito, noi siamo lo Stato, noi diamo ordini e i cittadini sono un gregge di pecore che deve obbedire e, se non obbedisce, viene sanzionato. Invece i cittadini andrebbero coinvolti, anche dal punto di vista della scelta delle decisioni da prendere, anche nell'immediato, quando si tratta di decisioni che comportano modifiche, persino gravose, alla loro vita privata. Coinvolgiamo i cittadini, signori. Noi non siamo quelli che stanno in alto e diciamo «fate così»: noi siamo quelli che dovrebbero fare in modo che la nostra popolazione si faccia partecipe di scelte che sono necessarie anche per lei. Lo dico senza intento polemico: è chiaro che certe dichiarazioni del ministro Musumeci non possono essere la cifra del modo con cui le istituzioni si interfacciano ai cittadini della zona. Ci vogliono un'altra sensibilità, un'altra trasparenza e rigore, perché altrimenti, giustamente, i cittadini se ne lamenteranno. Mi dispiace dover annunciare qui il mio voto di astensione. *(Applausi).*

Signora Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, anticipo il voto di astensione di Italia Viva-Il Centro-Renew Europe su questo provvedimento; astensione dovuta al fatto che, quando si tratta di salute e di tutela dei cittadini, noi non possiamo votare contro. Ma dire che questo decreto ci convince appieno

un provvedimento strutturale, visto che l'area dei Campi Flegrei è da 80.000 anni che vive momenti di terremoto e di bradisismo, per cui non è una realtà La realtà moderna forse è la maggiore sensibilità verso fenomeni che si stanno susseguendo, soprattutto in quest'anno, e che hanno creato un giusto allarme. È una zona unica per bellezza naturale e per bellezza archeologica, perché è frutto di una storia antica che risale ai tempi dei romani e che ci lascia delle pagine di bellezza straordinarie. Ci lascia anche, purtroppo, l'abusivismo degli anni Settanta e Ottanta, quando si è costruito in zone che oggettivamente non potevano essere considerate edificabili. Questo decreto nulla dice sull'argomento. Non c'è una norma che vieti le nuove costruzioni. Spero nel buon senso. Non si parla assolutamente di di riposizionare gli edifici altrove, pagina dolorosa e difficile, ma, se si parla di salute dei cittadini, forse dovrebbe essere il primo elemento. Si parla di capacità antisismica degli edifici, edifici che sono stati costruiti in zone dove non avrebbero dovuto essere costruiti dubito che potranno avere quell'autorizzazione da parte degli organi tecnici. Quindi, che valore avranno quegli immobili? In un colloquio informale con il ministro Musumeci c'è stato addirittura il tentativo di prevedere un'assicurazione obbligatoria per i cittadini; per fortuna non ha visto la nascita in questo provvedimento, perché dubito che le assicurazioni sarebbero corse ad assicurare edifici che sono stati costruiti in luoghi dove non dovevano sorgere.

lo Stato che centralizza tutte le competenze dei vari Ministeri all'interno della Presidenza del Consiglio e che dà quindi risposte rapide agli enti locali. Gli enti locali non hanno la forza di fare dei piani di evacuazione puntuali; la dovrebbe avere molto di più lo Stato, anche perché altrimenti si creano allarmismi e, quindi, anche resistenze da parte di chi deve lasciare quell'abitazione. Forse ci vuole l'autorevolezza dello Stato; non che gli enti locali non ce l'abbiano, ma magari lo Stato ha una maggiore forza nell'evitare di essere ricattabile da elezioni comunali che vedono il sindaco molto più vicino ai cittadini e molto più terzo nel dover dire loro di lasciare le proprie abitazioni. Soprattutto, avremmo voluto vedere il completamento di quelle infrastrutture che servono per un piano di sicurezza effettiva dei cittadini, come il famoso tunnel che dovrebbe essere autorizzato e consentire alle popolazioni di fuoriuscire a Pozzuoli che, nonostante le risorse e nonostante il suo semi-completamento - dico "semi" perché deve essere finito - deve essere ancora autorizzato. Questo però era un decreto-legge che serviva per l'emergenza. Se non è un'emergenza completare un'opera,

"per testimonianza", perché anche su un provvedimento del genere siete riusciti a fare un'unica lettura. Ed è veramente incredibile, perché nessuna forza politica ha fatto ostruzionismo su questo provvedimento *(Applausi)*, tanto un incontro politico - e lei c'era, Sottosegretario - con il ministro Musumeci per dichiarare - devo dire a nome di tutti i partiti - la più totale collaborazione su un provvedimento del genere. Si parla salute dei cittadini e di tutela delle vite e, quando si parla di questo, tendenzialmente anche le opposizioni riescono ad evitare di fare ostruzionismo. Nonostante questo, siete riusciti a fare un'unica lettura alla Camera e a non fare quegli approfondimenti secondo me

perché quei vulcani continuano a esistere e in quei paesi si continua a costruire, ci doveva essere una visione di prospettiva e non di emergenza.

Avete escluso luoghi in cui fenomeni tellurici ci sono; non abbiamo indicato dei luoghi che stanno in Trentino e che non vivono l'emergenza continua. Sono Comuni vicini vicini alla zona rossa che voi avete indicato e che ci chiedono: perché noi no? Non abbiamo presentato emendamenti perché volevamo essere pignoli, ma perché le comunità locali ci hanno detto che non si sentivano sicure Francamente, forse avrei fatto una riflessione di maggiore elasticità per la zona rossa, perché capisco che non bisognava creare allarmismo, ma abbiamo fatto un decreto emergenziale e d'urgenza e, se non bisognava fare allarmismo, allora dovevamo fare un provvedimento strutturale. Visto che abbiamo fatto un decreto d'emergenza vuol dire che c'è un'emergenza e vuol dire che le persone si sentono coinvolte in uno stato emergenziale. Se i cittadini chiedono di entrare nella zona rossa, sapendo tutto ciò che vuol dire, e cioè che le loro case saranno attenzionate e che il loro valore probabilmente verrà anche ridimensionato, vuol dire che hanno bisogno di avere quelle rassicurazioni che nemmeno in un ordine del giorno siete riusciti a dare.

ascoltiate i suggerimenti delle forze di opposizione, che in alcuni casi, come nella nostra, anche amministratori locali; abbiamo i consiglieri regionali, non siamo da un'altra parte, e probabilmente viviamo la realtà

per monitorare, ma anche per dare risposte immediate alle popolazioni e agli enti locali. Concludo. Il PNNR dimostra come

fattivamente la propria autorevolezza? Questo in collaborazione con la Regione e con gli enti locali - nessuno vuole fare un esproprio di competenze, ci mancherebbe - ma dando l'*imprimatur* che invece in questo provvedimento faccio fatica a vedere.

rispetto al fenomeno del bradisismo che da diversi mesi attraversa la zona dei Campi Flegrei, anche e soprattutto per cercare di venire incontro a tutta una serie di esigenze del territorio. I Campi Flegrei - ricordiamolo, soprattutto per chi ci ascolta e anche per lasciare una traccia agli atti - sono un'area vulcanica situata a ovest di Napoli che include alcuni Comuni importanti, come Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida, Quarto, Giugliano e anche una parte della città di Napoli. A differenza del Vesuvio, i Campi Flegrei non sono caratterizzati - come sappiamo - da un solo edificio vulcanico, ma sono invece un vero e proprio campo vulcanico attivo da circa 80.000 anni, con diversi centri vulcanici situati al centro e in prossimità di un'area depressa, che viene chiamata caldera. La caldera dei Campi Flegrei è soggetta a un lento movimento di sollevamento e di abbassamento del suolo che prende il nome di bradisismo. Durante il mese di agosto, nell'area dei Campi Flegrei l'Osservatorio ha registrato 1.118 terremoti; in particolare, nella notte fra il 26 e il 27 agosto si è registrata la scossa più forte in assoluto (4.2 di magnitudo), legata ovviamente all'innalzamento del suolo. Nonostante l'attività di monitoraggio dell'Osservatorio vesuviano, che naturalmente ringraziamo per il lavoro puntuale che svolge per la sicurezza del nostro territorio, con le strutture tecniche, nonostante anche le rassicurazioni riportate, evidentemente si è ingenerata una preoccupazione molto forte nella popolazione per questa intensa e continuata attività attività sismica. In generale, la densità degli abitanti, che pure è stata ricordata nel dibattito di oggi, e la particolare conformazione urbanistica

alla Camera, peraltro con il parere favorevole del Governo e del sottosegretario Freni che era presente alla seduta, fu votato un ordine del giorno fortemente voluto dal Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra

ritenendo che quello pensato fosse uno strumento necessario per uno specifico territorio e soprattutto che fosse indispensabile agire con prontezza per la messa in sicurezza degli edifici. passati dieci mesi da quel momento, ma purtroppo non si è dato seguito all'impegno preso. Oggi, in questo decreto-legge, manca un punto che noi riteniamo fondamentale, e cioè l'intervento sulla questione che più ci preoccupa, che è esattamente quella che riguarda l'edilizia privata. Questo decreto, infatti, prevede misure strutturali e misure di natura non strutturale; tra quelle che hanno caratteristiche maggiormente strutturali vi sono certamente il piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate e la verifica della funzionalità delle attuali infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali. Aggiungiamo che, in attuazione del decreto, è stata individuata la cosiddetta zona rossa per il rischio bradisismico, che coinvolge 85.000 persone e 15.000 edifici, che naturalmente sono concentrati prevalentemente nei Comuni di Pozzuoli e di Bacoli e in parte nella zona occidentale della Città metropolitana di Napoli. Tra le misure invece non strutturali, vi sono un piano di comunicazione alla popolazione, un piano speditivo di emergenza nell'ambito di una più alta pianificazione di protezione civile già in vigore e un potenziamento della risposta operativa territoriale di protezione civile. Vediamo però, oltre alle misure che sono previste, anche quello che dal nostro punto di vista manca, a partire dall'assenza di interventi per incentivare la messa in sicurezza degli edifici. Voglio aggiungere però a questo primo punto anche una seconda obiezione, perché credo che manchi, ancora una volta, anche in questo provvedimento, una parola chiara su uno dei grandi problemi che riguardano il nostro Paese, soprattutto con riferimento a quelle zone che sono più soggette o a rischio sismico o anche a rischio di dissesto idrogeologico,

Parlamento dotasse il nostro Paese di una legge contro il consumo del suolo che drammaticamente manca in Italia. Anche in questo caso, i dati dell'Ispra ci dicono

in pieno inverno demografico, ma - nonostante questo - alla riduzione demografica non corrisponde in alcun modo la riduzione del consumo di suolo. Vorrei dire che questo mi sembra un punto davvero essenziale. Il decreto - a nostro avviso - non risolve nemmeno il problema molto grave delle vie di fuga. Ci riferiamo a Comuni come quello di Pozzuoli, in cui si stimano circa 15.000 immobili residenziali; alla fine del 2021 la popolazione registrata in quel solo Comune era di 76.952 abitanti, nel 2011 superava gli 83.000. La Protezione civile per il momento ha verificato soltanto 4.000 edifici, relativi al 26 per cento della popolazione; e proprio mentre il bradisismo tra agosto e settembre accelerava la sua intensità, evidentemente queste scosse hanno messo in profondo allarme i residenti. Mi pare di poter dire che questi due fattori debbano essere davvero messi sotto esame: la stabilità degli edifici da una parte e le vie di fuga dall'altra. Molte zone controllate sorgono in grandi quartieri popolari, che peraltro sono stati anch'essi realizzati a seguito delle crisi bradisismiche del 1970 e del 1983. Chi di noi, come me, è napoletano e ha fatto politica a Napoli per tanti anni naturalmente ricorda perfettamente quello che sto dicendo. Dopo lo sciame del 1970, Pozzuoli venne sfollata, alcune aree della città come il rione Terra furono chiuse definitivamente. Negli anni Ottanta, quindi più recentemente, palazzi di epoca fascista in tufo, nella zona alta di Pozzuoli, vennero abbattuti perché pericolanti; i cittadini di queste due zone furono reindirizzati nei megaquartieri popolari del rione Toiano e di Monteruscello, mentre il resto della popolazione fece ritorno nelle vecchie abitazioni. Sui Campi Flegrei in un ventennio si è proceduto a una cementificazione del tutto slegata dall'edilizia precedente, sacrificando peraltro quella che era una vocazione agricola di terre fertilissime, che hanno una antichissima storia. Nei nuovi rioni sono stati realizzati dei grandi palazzoni, ma ci si è dimenticati delle vie di fuga commisurate a una popolazione totale addensata in circa 43 chilometri quadrati. Peraltro, nonostante il coordinamento dei sindaci dei Campi Flegrei con la Regione e con la Città metropolitana e nonostante il dialogo con il ministro Musumeci, che pure evidentemente ha rappresentato un elemento positivo, sulla questione specifica delle vie di fuga e in particolare sull'asse viario non si è - almeno a nostro avviso - intervenuti con la dovuta fermezza. Esiste un tunnel, una galleria, un collegamento veloce tra il parco urbano di Bagnoli e la tangenziale e la tangenziale di Napoli, che è costato 150 milioni di euro, i cui lavori sono determinati, ma che però non è ancora aperto perché il Comune non è in grado di pagare la manutenzione che costa 800.000 euro all'anno. conclusione, aggiungo semplicemente che proprio a riguardo della vicenda del tunnel è in atto una diatriba, perché il Comune vorrebbe - peraltro giustamente - che fosse la tangenziale di Napoli a prendere in gestione il tunnel, visto che si tratta di un'asse che collega la tangenziale di Napoli, gestita per l'appunto dall'ANAS, mentre la tangenziale di Napoli SpA non vuole prendere in gestione questo tunnel, o meglio lo prenderebbe in gestione soltanto a patto che fosse il Comune a pagare. dico che questo tunnel è evidentemente una via di fuga di fondamentale importanza e che sarebbe quindi assolutamente necessario capirlo. Aggiungo anche come elemento di riflessione che stiamo parlando di un asse viario, quello della tangenziale di Napoli, che è l'unico a pagamento in Europa da oltre quarant'anni.

del tunnel e della tangenziale e il fatto che non lo abbia fatto mi sembra un errore. Per queste ragioni annuncio il voto di astensione del Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra.

alle eruzioni vulcaniche da circa 80.000 anni e rappresentano quella che si definisce una grande caldera in stato di quiescenza. In epoca preistorica e protostorica era abitata da una popolazione tribale, nonostante l'intensità dell'attività vulcanica la rendesse in gran parte invivibile. I Campi Flegrei - come raccontano leggende, memorie e miti della storia - furono conosciuti per essere stati la sede del più importante porto di epoca romana, prima che venisse costruita Ostia, la piccola Roma, oggi meglio nota come Pozzuoli. I siti archeologici, i fenomeni vulcanici e la bellezza dei territori ne hanno fatto una località turistica tra le più visitate e sono un luogo talmente magico da venire persino cantato in tempi più recenti da Edoardo Bennato: «Campi Flegrei, gente che va; tempo d'aprile, qualche anno fa;

terreni vulcanici sono stati costruiti edifici e avviate attività imprenditoriali. Di recente ci sono state manifestazioni di vita di questo che è un vulcano, proprio sotto le case di una zona che va da Pozzuoli a Posillipo, per un diametro di circa 18 chilometri; il bradisismo che si è verificato ha ovviamente allarmato chi vive in quelle zone e noi tutti, anche perché eventi di bradisismo avevano modificato il territorio nel passato, tra il 1970 e il 1972 e poi tra il 1980 e il 1984, con addirittura 10.000 eventi sismici e un tasso di sollevamento del terreno di circa 180 centimetri. Già allora gli abitanti del rione Terra di Pozzuoli vennero evacuati e messi in sicurezza. Il Governo ha pensato che fosse giusto e doveroso intervenire con un decreto-legge, che certamente non può fermare il bradisismo ed eventualmente un'eruzione vulcanica, ma che introduce norme puntuali per monitorare ogni movimento dell'area vulcanica e per preparare un'eventuale evacuazione qualora l'attività bradisismica diventasse pericolosa per la popolazione. Innanzitutto, quindi, si tratta di un decreto-legge per rassicurare coloro che vivono sopra i Campi Flegrei che lo Stato c'è e si occupa di loro e del loro territorio; in secondo luogo, per riuscire, attraverso un monitoraggio più puntuale di quello che accade sotto terra, ciò che potrebbe accadere e, di conseguenza, valutare per tempo eventuali piani di sgombro. La gente di quelle zone vive e ha sempre vissuto in tranquillità, tanto che ci ha costruito e ci svolge le proprie attività. Anche se la Campania è nota al mondo per il Vesuvio e per quella grande eruzione che coprì la città di Pompei, che tutti vogliono visitare, l'area flegrea vede luoghi bellissimi, con un alto livello della qualità della vita, in cui vivono persone note per la cordialità e la simpatia. L'intervento normativo in esame mira proprio ad evitare eventi luttuosi, come quelli che hanno interessato la Campania, ad esempio a Ischia e Sarno. Si trattava di eventi di altra natura, ovviamente, ma sono stati avvenimenti luttuosi che forse, attraverso un intervento preventivo, avrebbero contato minori danni. Anche ad Ischia, per esempio, si sta provvedendo, oltre che a riparare quanto danneggiato dalla recente frana, a mettere in sicurezza il territorio contro nuovi danni da eventi alluvionali. Sono interventi che vengono portati avanti da un commissario nominato dal Governo, che contano su risorse adeguate: sono stati pianificati 181 interventi, di cui 61 conclusi e altri 28 cantierati. in esame prevede misure opportune, che hanno anche la puntuale copertura finanziaria per circa 53 milioni di euro. Innanzitutto, vi è uno studio di microzonazione sismica; si provvede, quindi, a un piano di rilevazione, che prevede un'analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata, ma anche a un piano per l'edilizia pubblica. Lo scopo è quello di individuare le misure più idonee di mitigazione, valutandone i costi. quindi un programma per l'implementazione del monitoraggio sismico e delle strutture. Saranno individuati i modi per delimitare la zona di intervento e gli eventuali piani di fuga. Il fine è quello di realizzare un piano di evacuazione che consenta a tutti gli abitanti di quell'area di porsi in salvo. Ovviamente contiamo sul lavoro prezioso che sarà affidato alla Protezione civile, che sarà in grado di individuare le soluzioni migliori. Sempre la Protezione civile, in accordo con la Regione Campania, dovrà realizzare il più opportuno piano di comunicazione a tutta la popolazione. Tutti gli abitanti, in particolare i soggetti più deboli, verranno messi a conoscenza dei rischi che corrono e le conseguenti procedure di emergenza, definite in un apposito piano, potranno essere adottate nel modo più opportuno. Tutte le procedure da adottare in caso di aggravamento del fenomeno bradisismico potranno essere adottate. Ovviamente noi contiamo sul pieno coinvolgimento delle realtà locali. poi importante verificare la funzionalità dei trasporti e di tutti i servizi essenziali, così come dovrà essere garantito l'accesso alla tangenziale di Napoli. il provvedimento individui puntualmente tutti i problemi da affrontare e da risolvere e ovviamente lo fa nel tempo necessario a mettere in piedi un'organizzazione complessa come quella immaginata per un evento che sarebbe epocale. La Campania e i suoi cittadini stanno facendo passi da gigante verso un'economia che cresce a passi da gigante, consentendo ai propri settori di competere con economie di altri distretti industriali, italiani ed esteri. Allo stesso modo, le istituzioni saranno in grado di dare prova di sé per intervenire in caso di emergenza in un eventuale evento - scusate il gioco di parole -augurandoci che i piani predisposti non debbano essere mai adottati. Per queste ragioni, i senatori di Forza Italia esprimeranno un voto favorevole sul provvedimento.

Signor Presidente, Sottosegretario, colleghi, colleghi, in questi giorni stiamo discutendo di una problematica che insiste sulla mia terra. Parliamo di un fenomeno che si accompagna al destino di centinaia di migliaia di concittadini, tra cui parenti stretti, amici, alcuni colleghi, tra l'altro presenti oggi in Aula. E allora, pur nella difficoltà di discutere atti che impatteranno sulla quotidianità presente e futura, non solo del popolo flegreo, ma di tutta la fascia interessata al fenomeno del bradisismo, il mio e il nostro contributo, quello del MoVimento 5 Stelle attraverso l'attività emendativa sia alla Camera che al Senato, è stato sempre orientato unicamente al miglioramento dell'Atto Senato 952, detto decreto Campi Flegrei. I meravigliosi Campi Flegrei, Presidente, che però con il fenomeno del bradisismo condizionano la vita dell'*hinterland* napoletano con epicentro nel comune di Pozzuoli. Il MoVimento 5 Stelle, con la rappresentanza dei parlamentari del luogo, tra i quali saluto e ringrazio l'onorevole Antonio Caso, per l'impegno profuso, ha posto sin dall'inizio della legislatura il tema del bradisismo a livello nazionale. Lo ha fatto con incontri istituzionali, ad esempio con il capo della protezione civile, l'ingegner Curcio, e il presidente dell'Istituto di geofisica e vulcanologia, il professor Doglioni. Il MoVimento 5 Stelle lo ha fatto invogliando i sindaci dei Comuni interessati e promuovendo un tavolo di lavoro tecnico sul fenomeno. Lo abbiamo fatto con attività legislativa vera e propria, attraverso ordini del giorno che sono stati approvati alla Camera. Lo abbiamo fatto altresì richiedendo audizioni continue sul tema. L'obiettivo, Presidente, è stato sempre lo stesso: mettere in campo tutte le azioni e le misure possibili per permettere ai cittadini di convivere con il fenomeno vulcanico e quello bradisismico, facendolo nella massima tranquillità possibile per salvaguardare l'incolumità delle persone, ma allo stesso tempo anche il tessuto sociale ed economico del territorio. Parliamo di un'area dove insistono la vita, i sogni, gli investimenti e le aspirazioni di oltre 500.000 persone;

Presidente, proviamo ad immaginare lo stress di queste persone, di cui però si rende complice anche una comunicazione inadeguata come quella dell'ultima relazione della Commissione grandi rischi dello scorso mese che ha indotto il ministro Musumeci ad ipotizzare l'ingresso nell'allerta arancione, per poi fare dietrofront dopo una settimana. una settimana. Per i cittadini flegrei quella settimana è stata un inferno. Sapete infatti cosa significa passare in allerta arancione? Significa che vengono svuotati gli ospedali, le case di cura, le carceri, la popolazione è invitata ad allontanarsi con un contributo statale in aree lontane e l'economia complessiva di un'area è annullata. Insomma significa la distruzione di un tessuto urbano, economico e sociale.

abbiamo lavorato con senso di responsabilità ed elevata empatia, evitando qualsiasi strumentalizzazione o giochi politici. Lo abbiamo fatto anche ieri in Commissione, fino all'ultimo minuto, con i nostri emendamenti ed ordini del giorno.

su cui lavorare perché troppi sono ancora gli elementi lasciati in sospeso e le domande a cui non si è data risposta. Riteniamo, per esempio, che sia miope la visione di lasciare che l'impianto base del decreto-legge si occupi esclusivamente degli effetti sismici del bradisismo e poco o nulla della prevenzione e della mitigazione del rischio vulcanico. Nell'ottica della nostra massima collaborazione,

perfino a quelli di essi non onerosi. Governo e maggioranza, signor Presidente, hanno detto di no al sismabonus e al potenziamento della rete di monitoraggio e dell'aumento di personale dell'Osservatorio vesuviano; agli aggiornamenti dei piani di emergenza vulcanica e al miglioramento delle vie di fuga per tutti i Comuni della zona rossa; zona rossa; all'analisi di vulnerabilità e al consolidamento del patrimonio archeologico; a un osservatorio permanente per il monitoraggio strutturale di edifici e infrastrutture. Mi lasci dire, signor Presidente, che di certo non aiuta leggere in una nota stampa il ministro Musumeci affermare che sui Campi Flegrei non si presta a strumentalizzazioni e preferisce non ascoltare le voci delle opposizioni, né quelle della maggioranza, ma obbedisce solo alle esigenze del territorio. Beh, signor Presidente, questo non ha reso assolutamente facile il nostro lavoro, però vorrei innanzi tutto ricordare al Ministro che, fino a prova contraria, deve rispondere al Parlamento. Quanto poi alle esigenze del territorio, allora posso benissimo esporle io al signor Ministro, perché le domande sono state tutte evase con la nostra attività emendativa, ma sono state respinte interamente e - badate bene, signor Presidente - per partito preso. Questa è una constatazione di fatto, da non confondere con una polemica. In che modo poi avremmo mai potuto strumentalizzare questo provvedimento? Noi quelle scosse le avvertiamo le viviamo con angoscia sulla nostra pelle, quindi l'ultima cosa che ci verrebbe in mente di fare, signor Presidente, è un uso strumentale della vicenda per vantaggi politici.

e non con la solita procedura d'urgenza con cui si prova a svuotare il mare con le mani, sprecando anche le poche risorse messe a disposizione. Insomma, signor Presidente, se abbiamo a cuore il destino degli italiani, di tutti gli italiani,

come quella del governatore campano e commissario straordinario De Luca, per il quale i fondi stanziati sarebbero del tutto insufficienti, credo si tratti invece del primo provvedimento in tema di prevenzione del rischio sismico legato al bradisisma dei Campi Flegrei addirittura dal 1984. quarant'anni e non si è mai intervenuto con misure specifiche aggiuntive o aggiornate per tentare di mettere al riparo la popolazione di quell'area dal rischio incombente a causa dell'attività vulcanica che la interessa. Già solo questo dimostra e fa capire ancora una volta quanto questo

anziché considerare insufficienti i finanziamenti messi in campo, bisognerebbe piuttosto gioire per la solerzia con cui ci si è attivati di fronte a questa emergenza e, casomai, lavorare insieme per migliorare quello che è migliorabile, come nel caso dell'apertura di nuove vie di fuga previste per esempio a Pozzuoli, grazie a un emendamento della Lega presentato D'altronde, 55 milioni di euro di risorse investite da un Governo che è al lavoro solo da un anno, dopo che i precedenti, compreso quello guidato dal presidente Conte, non avevano investito neanche un centesimo, sono la più chiara e puntuale testimonianza

Prevenzione è anzi la parola chiave di questo decreto, che ha l'enorme pregio di coinvolgere, a diversi livelli, tutti gli enti interessati, creando una sorta di filiera nella loro azione. Vengono infatti innanzitutto identificati quelli a cui è affidato il compito di studiare la situazione geologica. la predisposizione e l'attuazione di un piano straordinario, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, e sono previsti i lavori di delimitazione del territorio interessato, affiancando al Dipartimento della protezione civile una struttura di supporto tra esperti, amministratori locali e strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato. Vi è poi un'altra misura particolarmente importante e di rottura con il passato: il potenziamento e il ruolo centrale della comunicazione alla popolazione, per la quale sarà responsabile la Regione, sempre in raccordo con il Dipartimento della protezione civile e servendosi del contributo dei centri di competenza indicati nel decreto stesso, che hanno anche il compito di coordinare le attività. attività consistono nell'approvazione, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, di un piano di iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza dei rischi e delle buone pratiche di protezione civile, come ad esempio iniziative specifiche previste all'interno delle scuole delle delle aree interessate, incontri pubblici con la popolazione, corsi di formazione continua addirittura rivolti anche ai giornalisti dell'area, in modo che possano poi promuovere una migliore informazione al pubblico sul rischio e sulla pianificazione. poi l'installazione sul territorio della segnaletica. Un'ulteriore previsione che denota una grande sensibilità del Governo è quella di specifiche forme di comunicazione dedicate alle persone con disabilità. Prevedere quindi le migliori attività di prevenzione e di corretta e completa sensibilizzazione della popolazione perché sia consapevole dei rischi e sappia esattamente come muoversi in caso di necessità era quanto il Governo poteva e doveva fare ed è quanto ha fatto, con grande responsabilità e lungimiranza, andando poi anche a coinvolgere i Comuni interessati della zona rossa. Innanzitutto la città metropolitana di Napoli, che avrà un un ruolo di coordinamento di tutta una serie di attività, come la ricognizione dei fabbisogni urgenti ai fini del reclutamento del personale per potenziare la struttura comunale di protezione civile o l'allestimento di aree e strutture temporanee per accogliere la popolazione, anche al di fuori del proprio territorio e in deroga alle destinazioni d'uso degli strumenti urbanistici, e che dovrà attivare, per esempio, procedure straordinarie per gli appalti pubblici in caso di somma urgenza. Anche in questo caso e sempre in linea con lo spirito che anima l'intera politica governativa, finalizzata a garantire l'interesse pubblico sburocratizzando tutti gli *iter* amministrativi, si prevede infatti il ricorso a procedure semplificate e ad altre disposizioni di accelerazione proprio perché ogni intervento possa essere più rapido ed efficace, come la situazione richiede. È corretto anche richiedere la rendicontazione dei finanziamenti ricevuti dal governatore De Luca in qualità di commissario straordinario, per capire quanto e come siano stati spesi i soldi dello Stato finalizzati alla messa in sicurezza dell'area dei Campi Flegrei e da questo quadro poi capire come si possa dare un ulteriore contributo, magari individuando misure di accelerazione e semplificazione. È infatti chiaro che, nonostante il notevole sforzo fatto da questo Governo, questo è anche per noi solo un primo passo verso l'obiettivo, a cui ne seguiranno altri (voglio rassicurare il senatore Nava), così come è stato ad esempio anche per Ischia, per restare sempre in zona di territorio campano. campano. Il percorso - lo sottolineo ancora - è iniziato finalmente, dopo decenni d'inerzia, e andrà avanti su questo solco, che ci sembra assolutamente positivo e propositivo. Per questo, a nome del Gruppo Lega, dichiaro il nostro convinto voto favorevole. Presidente, colleghe e colleghi, siamo chiamati oggi a convertire un altro decreto-legge, con gli ormai consueti tempi strizzati di un monocameralismo alternato, prassi ormai tristemente consolidata. una distorsione che abbiamo provato già a denunciare e che, ancora una volta e in questo caso ancor di più, ci invita a riflettere, considerando soprattutto che questo provvedimento interviene su una situazione delicata, quella dell'area dei Campi Flegrei, che non pone solo questioni di carattere emergenziale, ma si lega anche a caratteristiche strutturali di quel territorio e del suo tessuto urbanistico e sociale. Proprio per questo, se il decreto-legge è, almeno in questo caso, strumento appropriato, concentrare la discussione in una sola Camera, che pure ha fatto - va riconosciuto - un lavoro di miglioramento importante del testo, continua a porre problemi che quest'Aula credo non possa e non debba ignorare. Nel corso degli ultimi mesi, come già detto da molti dei colleghi che mi hanno preceduto, nell'area flegrea si sono verificati oltre mille eventi sismici, il più significativo dei quali - lo hanno ricordato tutti - ha raggiunto magnitudo 4.2. L'intensificarsi del bradisismo e il rischio solo in parte - ricordiamolo - connesso di fenomeni eruttivi hanno comprensibilmente gettato nel panico la popolazione dei Comuni di quell'area. Si tratta di Comuni che, come noto, sono intensamente popolati, altrettanto intensamente - ahimè - edificati e che, come altrettanto noto, soffrono importanti carenze infrastrutturali, soprattutto con riferimento ai trasporti e dunque alle vie di fuga e alla concreta possibilità di articolare piani di evacuazione realmente efficaci. Mentre si svolgevano i lavori della Camera, la Commissione grandi rischi ha evidenziato, anche a seguito di approfondimenti tecnici sul bradisismo in atto, numerose criticità legate all'aumento della pressione sotterranea e all'aumento della concentrazione dei gas nelle fumarole, non potendo escludere il verificarsi di esplosioni freatiche nel sistema Solfatara-Pisciarelli, nonché, più in generale, di un ulteriore aumento della sismicità, così come di fratture superficiali e risalita di magma in un arco temporale che va da alcuni mesi a pochi anni.

previsti dalla pianificazione di emergenza vulcanica». Infine, ha raccomandato un'intensificazione delle attività di monitoraggio e delle attività di prevenzione in preparazione all'eventuale necessità di passare rapidamente verso un livello di allerta superiore. Le affermazioni della Commissione grandi rischi sono state al centro delle preoccupazioni dei colleghi della Camera, che ne hanno tenuto conto nel lavoro di miglioramento del testo del decreto-legge. Un miglioramento che va riconosciuto, che indubbiamente c'è stato, ma che purtroppo non ha risolto tutte le criticità evidenziate soprattutto da chi, come i sindaci dell'area e i rappresentanti dell'ANCI, hanno sollevato il problema e di cui il Partito Democratico e tutte, a dir la verità, le forze di opposizione si sono fatti responsabilmente carico in questa discussione. Il decreto-legge, anche grazie alle modifiche apportate alla Camera, rappresenta indubbiamente un passo in avanti nella gestione dell'emergenza di quell'area. Permangono però, come pure abbiamo sottolineato in tanti, troppe criticità che non sono solo puntuali, ma esprimono un difetto sistemico, direi, nell'approccio al problema.

con comprensibile urgenza, certo, e altrettanto comprensibile difficoltà di reperire tutte le risorse adeguate. Il decreto-legge, infatti, stanzia circa 50 milioni di euro a copertura degli interventi previsti, ma lo fa per un periodo di tempo molto limitato, cioè anni 2023-2024. L'approccio rimane solo quello di tamponare l'emergenza, senza preoccuparsi di creare in alcun modo le condizioni perché quell'emergenza non si riproponga più. Lo abbiamo osservato tante volte in quest'Aula; io stessa ho avuto modo di dirlo, per esempio quando ci siamo occupati della vicenda Ischia. Ricordiamolo ancora una volta: il modo migliore per affrontare le emergenze è evitare che si verifichino ancora. Evitare, cioè, che per le specifiche caratteristiche di un territorio e del suo tessuto urbanistico e sociale, eventi naturali imprevedibili, ma, come nel caso dell'area flegrea, connaturati anche alla storia e alla conformazione di quel territorio, producano emergenza. su questo nel decreto-legge si fanno passi in avanti, ma non sufficienti. Guardiamo però adesso al bicchiere mezzo pieno. Facciamo riferimento in particolare all'articolo 2, che disciplina - come hanno detto già tanti - il piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico; e all'articolo 3 che, grazie anche all'azione del Partito Democratico, disciplina il piano di comunicazione alla popolazione da attuare in raccordo con i Comuni della zona rossa. L'intervento però, come dicevamo, si ferma qui. Il problema viene individuato, le criticità vengono comunicate alla popolazione e mi verrebbe da dire: poi cosa facciamo? Nulla si prevede soprattutto in chiave pluriennale e sistemica per mettere quei Comuni e le popolazioni interessate nelle condizioni di attrezzarsi per rafforzare la prevenzione. Non ci sono infatti risorse pluriennali per mettere in sicurezza gli edifici, eppure le avevamo chiesti a gran voce; e non ci sono misure di sostegno e di finanziamento degli interventi privati di consolidamento e messa in sicurezza, come pure avevano chiesto in tanti. Penso per esempio all'istituzione del super sismabonus chiesto da tanti sindaci e, non ultima, dall'ANCI. Nemmeno è stata raccolta, come pure è stato già ricordato, la proposta delle opposizioni di equiparare l'area flegrea a zona sismica 1, ossia ad elevata pericolosità, il che avrebbe consentito di attivare, per esempio, una serie di importanti dispositivi di prevenzione e gestione di eventuali emergenze. Un miglioramento si è avuto sulle possibilità di assumere personale specializzato da parte dei Comuni: anche questo è già stato ricordato. Era previsto che ciò potesse accadere inizialmente per dodici mesi; siamo arrivati a ventiquattro, ma - ricordiamolo - la richiesta dei Comuni, non a caso, era di trentasei mesi, ovviamente per avere il tempo di pianificare interventi necessari interventi necessari con la dovuta professionalità. Una richiesta che, a dir la verità, mi pareva semplicemente, oltre che condivisibile, di buon senso. Eppure anche questa non è andata in porto. Importanti questioni aperte sono poi quelle relative al miglioramento dell'infrastruttura viaria e del trasporto intermodale. Chi conosce quei territori - sono campana e napoletana, come molti di coloro che sono intervenuti questa mattina sa benissimo che si tratta di aree fortemente popolate e difficilmente evacuabili in assenza di vie di fuga ben organizzate. Non a caso, la questione proprio delle vie di fuga era già stata al centro della legge n. 887 del 1984, adottata in occasione dell'ultimo importante fenomeno bradisismico. Nella legge citata ci sono interventi non ancora attuati o non del tutto. Anche qui avevamo chiesto di dare priorità alla loro conclusione; la richiesta è stata accolta soltanto in parte. L'esempio del tunnel, pure riportato da tanti, che collega il porto di Pozzuoli alla tangenziale di Napoli è cruciale: un tunnel di 1.100 metri già pronto e tuttavia non ancora aperto al transito. Questo perché il Comune non ha risorse sufficienti per la sua gestione e manutenzione. Alla Camera se n'è discusso molto e abbiamo ottenuto almeno che tale opera venisse espressamente menzionata nel testo del decreto-legge, dando la possibilità al Comune di Pozzuoli di avvalersi di Anas SpA, anche sulla base di una specifica convenzione: di nuovo un passo in avanti, ma ancora una volta un passo a metà; un passo in avanti ancora nella logica dell'emergenza e senza un vero ragionamento di prospettiva. Avevamo chiesto di coinvolgere stabilmente nella gestione del tunnel la società che si occupa della tangenziale di Napoli, perché si trattava di un'asse viario servente rispetto a quell'arteria. Questo avrebbe dato sicuramente maggiore certezza, anche perché vi erano già interlocuzioni importanti in questo senso tra i soggetti interessati. Tutte le richieste di modifica che ho ricordato sono state riproposte dal Partito Democratico in Commissione anche qui al Senato, a dimostrazione del fatto che per noi resta fondamentale l'adozione di una prospettiva sistemica e di lungo periodo nella disciplina di tutte le attività di prevenzione, di controllo e di gestione dell'emergenza. 50 milioni in nemmeno due anni sono insufficienti e restringono il campo d'azione rispetto a una situazione che, come ricordato dalla Commissione grandi rischi, è purtroppo assolutamente precaria. Ho voluto fare questi esempi non per mettere in dubbio l'importanza del lavoro fatto alla Camera, men che meno per piantare bandierine; non l'abbiamo mai fatto e non intendiamo farlo, soprattutto in una materia così delicata che deve essere affrontata con lo sforzo corale di tutte le forze politiche. L'ho fatto però per mettere in luce ancora una volta un limite strutturale nell'approccio alle emergenze. Le emergenze non sono mai naturali né inevitabili; le emergenze sono la conseguenza di un errore che si fa a monte nella gestione della relazione tra natura e attività umane. I Comuni e le popolazioni dell'area flegrea sanno benissimo cosa significa convivere con uno dei sistemi vulcanici più ampi ed estesi del mondo. Parliamo di 550.000 persone in un territorio caratterizzato da un tessuto urbanistico, edilizio e sociale davvero assai complesso. In un caso come questo, bisogna fare di tutto per evitare che eventi naturali estremi divengano emergenze. Questo e solo questo è stato lo spirito che ha guidato il Partito Democratico lungo tutta la discussione relativa al disegno di legge che oggi approviamo. Il dialogo - lo ricordo, infine - è stato ancora una volta franco e i miglioramenti ci sono stati, ma ancora insufficienti. Per questo, ovviamente, per il senso di responsabilità che è proprio del PD e con la responsabilità che è sempre necessario assumersi di fronte a una situazione tanto delicata, annuncio il voto di astensione del Gruppo Partito Democratico.

troppe volte quest'oggi anche in quest'Aula, non solo alla Camera dei deputati, è risuonata una parola orrenda, orribile, orrorifica: la parola «astensione».

perché dinanzi a provvedimenti come quello che stiamo andando ad approvare la logica dell'appartenenza dovrebbe cedere sempre il passo all'etica della responsabilità. Uno dei più grandi strateghi militari di tutti i tempi, Sun Tzu, diceva che la vittoria è possibile anche nelle battaglie più ardue quando soggetti diversi sono animati dallo stesso spirito e dinanzi a calamità, morti, distruzioni, sofferenze, ansie, stupisce, anzi mortifica la non scelta dell'astensione. E per questo fino all'ultimo in Commissione e in Aula abbiamo sperato in un ripensamento, in un ravvedimento operoso, in un sussulto di dignità dell'Assemblea.

sofferenza, addirittura. Quest'oggi le opposizioni hanno perso la grande occasione di dimostrare dalla opposizione di avere cultura di Governo, hanno smarrito il senso della responsabilità e mentre noi abbiamo deciso di decidere, loro hanno scelto di non scegliere e si sono rifugiati in un angolo di irresponsabilità. *(Applausi)*. La scelta di astenersi su un disegno di legge così delicato come quello sui Campi Flegrei, che per la prima volta affronta in modo organico, strutturato, coraggioso un problema epocale come quello del bradisismo (il sisma lento), ha il tanfo - consentitemelo almeno - a tratti

Von Clausewitz, diceva che il coraggio è di due tipi: quello fisico dinanzi al pericolo personale e quello morale dinanzi alle responsabilità. Queste responsabilità voi non avete voluto

dei sindaci del territorio, tutti, di sinistra o di centrosinistra, perché noi conosciamo il valore della collaborazione istituzionale.

Lo abbiamo fatto in primo luogo - e di questo ringraziamo il signor Ministro - con la tempestività e la immediatezza dell'intervento, con l'adeguatezza tecnica nella istruttoria che abbiamo svolto, con l'assunzione della responsabilità politica nelle decisioni che abbiamo assunto, naturalmente anche con la praticabilità delle soluzioni operative, con la sostenibilità finanziaria degli interventi che abbiamo posto in essere. con la connotazione strutturale, destinata quindi a prolungare l'impegno nel tempo, in una visione d'insieme che si chiama coerenza, che consente di armonizzare questo disegno di legge rispetto a tutti gli altri interventi che riguardano

che, ancor prima che da Bennato, sono stati cantati da Omero, che diceva che in quella pianura Giove aveva convocato gli dei dell'Olimpo per mortificare e distruggere i giganti. È la terra dove è approdato l'apostolo Paolo dopo la morte di Cristo; è la terra, per dirla con Madame de Staël, che è una porzione dell'universo in cui più che altrove vulcani, storia e poesia hanno lasciato il segno. Noi quel territorio abbiamo l'esigenza di proteggerlo, perché il bradisismo, un fenomeno epocale che naturalmente non possiamo ingabbiare, sta da millenni minando la sicurezza di quei territori con movimenti continui di innalzamento ed abbassamento del terreno. Lei, signor Ministro, ci ha onorato della sua presenza più volte nei Campi Flegrei e ricordo che con lei abbiamo visto insieme il tempio di Serapide, che non è mai stato un tempio romano, ma era il vecchio mercato al centro di Pozzuoli, dove c'è il primo rilevatore geologico della storia, le colonne ancora erette sulla cui superficie ci sono dei fori creati dai molluschi marini (quelli dello spazio intertidale),

vengano, quindi, signor Ministro, uno stanziamento coraggioso di 55 milioni di euro, un piano straordinario di studio della vulnerabilità sismica, un piano di mitigazione dei rischi, un piano di riqualificazione sismica sia per l'edilizia privata che per quella pubblica, un piano speditivo di emergenza, finalmente attività esercitative da parte del Servizio nazionale della Protezione civile. finalmente, il potenziamento della risposta operativa territoriale e, non da ultimo (perché non si è mai provveduto in questo senso), un piano trasparente e coraggioso di comunicazione alla popolazione interessata. Signor Ministro, siccome non abbiamo mai avuto paura delle parole, dico che questo è un intervento straordinario, perché grazie all'azione del Governo Meloni e grazie al coraggio e alla risposta

Per tacere, poi, per amore e per carità di patria del confronto con la palese, drammatica inadeguatezza della politica regionale, di un governatore che è ancora lì nonostante il Partito Democratico e che da otto anni è commissario straordinario di Governo, aduso soltanto alla sistematica manipolazione della realtà, immobile nelle sue responsabilità, incapace di fornire risposte, avvolto e sorretto insieme da una ragnatela ignobile di interessi e di clientele.

Signor Presidente, naturalmente mi assumo la responsabilità di quello che dico. Prima Ischia, poi Caivano, poi i Campi Flegrei: stiamo trasformando territori critici in modelli di riscatto, di amministrazione del territorio, di visione. Non vi seguiremo nel torbido angolo della convenienza politica o sull'altare della viltà, perché - e lo diceva Seneca - «non è perché le cose sono difficili che non osiamo; è proprio perché non osiamo che le cose sono difficili». Noi abbiamo il coraggio, il dovere, la volontà di decidere, signor Ministro, e per questo, con grande convinzione, annunciamo il voto favorevole di Fratelli d'Italia.

recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili***

Senatrice Nocco, la interrompo un attimo. Colleghi del PD, per cortesia: è da questo lato che proviene il rumore maggiore. NOCCO, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. Desidero innanzitutto ringraziare il presidente di Commissione, senatore Calandrini, e il rappresentante di Governo che ha partecipato alle sedute in Commissione, i correlatori, i colleghi Damiani e Borghi, e tutti i componenti delle Commissioni per il lungo lavoro svolto per migliorare il testo. Il provvedimento, all'articolo 1, reca una norma transitoria in materia di indicizzazione dei trattamenti pensionistici. Esso prevede l'anticipo al primo gennaio 2024 e al primo dicembre 2023 della decorrenza del conguaglio concernente il calcolo della perequazione relativa al 2022, con il ricalcolo in via retroattiva dei ratei di pensioni decorrenti dalla medesima data del primo gennaio 2023. L'articolo 1-*bis*, introdotto durante l'esame al Senato, reca disposizioni dirette ad armonizzare i trattamenti economici e accessori del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'ANPAL e dell'Agenzia italiana per la gioventù. L'articolo 2 differisce al 31 dicembre 2024 il termine per la trasmissione della richiesta di recupero da parte dell'INPS delle prestazioni pensionistiche indebite, con riferimento agli indebiti che emergano dalle verifiche dei redditi concernenti il periodo di imposta 2021, nonché agli indebiti che emergano dalle verifiche dei redditi relativi al periodo di imposta 2020, limitatamente alle verifiche in base ai dati trasmessi dal titolare del trattamento pensionistico e non già disponibili per una qualsiasi amministrazione pubblica. L'articolo 2-*bis*, introdotto in sede referente, attribuisce agli organismi di autoregolamentazione la facoltà di istituire una banca dati informatica centralizzata dei documenti; dati e informazioni che i professionisti acquisiscono nello svolgimento della propria attività professionale e che sono tenuti a conservare al fine di prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. L'articolo 3, commi da 1 a 3, dispone in via eccezionale per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle amministrazioni statali, un incremento a valere sul 2024 dell'indennità di vacanza contrattuale riferita al mese di dicembre 2023. dell'articolo 3, inseriti in sede referente, modificano la disciplina sul criterio di quantificazione al fine dell'inclusione nel computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente o nel computo dei redditi imponibili, equiparati o assimilati a quelli del lavoro dipendente, del beneficio relativo alle concessioni di prestiti. L'articolo 3, inserito sempre in sede referente, amplia una fattispecie transitoria, la quale consente fino al 31 dicembre 2026, in deroga alla normativa vigente, il conferimento di alcuni incarichi a titolo oneroso a soggetti già collocati in quiescenza. L'articolo 4, come modificato in sede referente, rinvia, per il solo periodo di imposta 2023, il versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL da parte delle persone fisiche titolari di partita IVA, che nel periodo di imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro. L'articolo 4-*ter*, inserito in sede referente, estende le esenzioni IVA per le prestazioni sanitarie anche alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona, volte a diagnosticare o curare malattie problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute anche psicofisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica. L'articolo 4-*quater*, introdotto in sede referente, abroga l'obbligo previsto a decorrere dal periodo di imposta 2023, per i sostituti di imposta che prestano assistenza fiscale,

delle fatture elettroniche emesse nei loro confronti. La norma infine introduce una semplificazione nelle modalità di espressione del parere conforme da parte dell'Agenzia delle entrate nei casi di proposta di transazione su crediti, tributi e contributi. Signor Presidente, rinnovo il mio ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato ai lavori e ringrazio anche per avermi concesso la possibilità di esporre la relazione.

ulteriore riflessione sul cosiddetto decreto anticipi, che inizia tutto il periodo delle due settimane che ci separano dalla dalla manovra finanziaria, che quest'anno vede il suo passaggio in prima lettura qui al Senato. Il decreto-legge in esame si chiama anticipi non soltanto perché anticipa la manovra finanziaria, ma anche e soprattutto perché

Inoltre, sono stati previsti anche 2,5 miliardi da dedicare al rinvio della seconda rata dell'anticipo delle imposte dei redditi dei titolari di partita IVA con dichiarazioni dei redditi sotto i 170.000 euro. Sono stati prorogati al 30 luglio i termini previsti per la regolazione delle sanzioni

Sono stati stanziati quasi 100 milioni di euro per gli alloggi e le residenze universitarie. C'è l'anticipo di un miliardo di euro per Rete ferroviaria italiana per continuare a sbloccare importanti opere infrastrutturali del nostro Paese. La nuova Sabatini è stata rifinanziata con altri 50 milioni di euro.

di coerenza di temi, è stato trattato in Commissione bilancio in modo prodromico alla futura trattazione del disegno di legge di bilancio, che è tuttora in corso.

in Commissione vanno secondo me nella direzione giusta, tant'è vero che c'è stato un clima che oserei definire *bipartisan* per buona parte della trattazione. Diciamo che il merito della Diciamo che il merito della realizzazione finale di questo testo è sicuramente da condividere con i colleghi dell'opposizione e penso che questo sia un buon modello da seguire. Ci sono alcuni punti Ci sono alcuni punti su cui vorrei soffermarmi. Il primo riguarda l'articolo 1, vale a dire l'anticipo dell'indicizzazione della perequazione delle pensioni. Stiamo parlando di pochi mesi, però il punto secondo me è importante, perché rileva l'attenzione che tutte le forze del Parlamento rivolgono ai pensionati, che sono ovviamente, così come i lavoratori dipendenti, i più danneggiati dall'inflazione. Un mese di anticipo in più, prima del Natale, sembra magari una piccola cosa, ma in realtà può aiutare tanta gente, tenuto presente che, quando si parla di pensioni, la platea è così ampia che bisogna muoversi con prudenza sulle cifre, perché è ovvio che anche piccoli cambiamenti e piccoli anticipi, seppur dovuti, comportano degli impegni importanti. In questo caso il decreto al Così come vorrei far notare, fra le aggiunte che ci sono state all'interno della trattazione, l'introduzione dei fondi di garanzia per le piccole e medie imprese,

cose che vanno in automatico, ma purtroppo non è così. Lo Stato deve stare attento: ogni volta che realizza una grande opera non finisce lì. Tante volte si pensa che la realizzazione dell'opera sia fine a se stessa. Non è vero. La grande opera continua a dispiegare i suoi effetti benefici; abbiamo visto, con le ultime ondate di maltempo, cosa sarebbe successo a Venezia se non ci fosse stata quest'opera, che però deve essere manutenuta. In questo caso si garantisce la possibilità della manutenzione del MOSE. Vorrei ricordare, sempre fra gli articoli introdotti, l'articolo 8-*quinques*. Anche in questo caso si parla di cose magari sembrano tecniche, ma la possibilità per i risparmiatori di avere più piani di risparmio, i cosiddetti PIR, in realtà rappresenta un passo avanti e sicuramente la possibilità per tanti di loro di avere una detassazione importante sui propri investimenti e al contempo allocare una parte maggiore dei propri investimenti rispetto a quello che c'era prima in attività produttive domestiche, con beneficio per l'economia in generale. Infine, vorrei porre l'accento su un emendamento importante che è stato gestito, secondo me, con estrema responsabilità da tutti i Gruppi, che è l'emendamento 14-*bis* relativo alla Strada dei Parchi, ricorderete - era stata oggetto di un esproprio di concessione da parte del Governo precedente. Evidentemente, ogni tanto qualcuno, quando è al Governo, si dimentica che ci sono dei limiti anche all'attività di arbitrio che può avere e in questo caso si era di fronte a un contenzioso che non si sa quanto sarebbe durato. Quando cominciano a scontrarsi diverse ragioni, si entra in un meccanismo che probabilmente non fa bene né allo Stato né alla parte in causa, vale a dire l'attuale concessionario dell'autostrada. In questo caso si arriva a una transazione onorevole che chiude la questione e che invece

argomenti che possono essere più o meno interessanti per buona parte dei cittadini, ma che in questo periodo

presenti in Parlamento, di dare un minimo di attenzione a quante più persone possibile per cercare di rendere la loro vita più semplice.

abbiamo finalmente superato una barriera che pesava ingiustamente su oltre 2.200 validi e giovani professionisti della nostra Nazione. Questi professionisti hanno lungamente sopportato un'ingiustizia. Colleghi, vi chiedo di lasciare liberi i banchi del Governo. Capisco una brevissima consultazione, visto che ci sono anche emendamenti in corso di valutazione, *(FI-BP-PPE)*. Questi professionisti hanno lungamente sopportato un'ingiustizia intollerabile: l'impossibilità di depositare i bilanci e di iscrivere atti societari nel registro delle imprese, nonché di iscrivere documentazione amministrativa mediante la trasmissione telematica degli stessi; un diritto che era garantito ad altri, ma negato a loro. Questo emendamento, firmato con il collega Lotito, non solo corregge un'ingiustizia storica, ma si allinea perfettamente con gli sviluppi contemporanei del nostro settore. Si inserisce in un contesto di aggiornamenti professionali e di transizione verso procedure telematiche più efficienti, conferendo a questi professionisti la piena agibilità delle loro competenze tecniche, riconosciute dalla legge, e permettendo loro di partecipare pienamente al processo di digitalizzazione dell'informazione aziendale. Forza Italia si conferma quindi ancora una volta al fianco dei professionisti, nella consapevolezza della loro importanza per la crescita e lo sviluppo del Paese. Questo è un passaggio importante, fondamentale, non solo per la semplificazione delle procedure, ma anche per l'edificazione di un sistema fiscale più equo e trasparente. Più che una semplice correzione di un testo di legge, questo emendamento elimina un paradosso che ha creato significative difficoltà sia per i diretti interessati sia per le imprese che si affidano alle loro *expertise*. Con questo gesto di giustizia ed equità dimostriamo che la nostra maggioranza di Governo non solo ascolta, ma agisce in risposta alle esigenze dei professionisti, favorendo un rapporto più efficace e collaborativo tra l'amministrazione finanziaria dello Stato e i contribuenti. L'approvazione di questo emendamento rappresenta un passo importante e necessario per sostenere i nostri professionisti nel ruolo cruciale di assistenza alle imprese. In un'era dominata dalla digitalizzazione e dalla necessità di trasparenza, facilitiamo un passaggio più fluido e integrato nel registro delle imprese, aumentando la fiducia e l'efficienza nel nostro sistema economico.

che ha inficiato negativamente anche l'economia tutta. Si è sempre fatto l'errore di sovraccaricare questa materia di troppe e sbagliate aspettative. Ciò ha portato nella direzione sbagliata e ha contribuito a perdere di vista le questioni più serie, la principale delle quali in materia forse è questa: come è possibile favorire l'occupazione? La risposta più ragionevole è che, a tal fine, occorre un rilancio economico che determini la creazione di posti di lavoro; prima di distribuire la ricchezza la si deve creare. È per questo che il nostro Governo, sin dal primo giorno, non ha pensato di dare risposte ritoccando qualche comma e dando nomi altisonanti ai decreti. Quanti ne abbiamo sentiti in questi anni con roboanti termini inglesi che nascondevano il nulla cosmico? Le risposte, lo sappiamo, sono altre e stiamo provando a darle: incremento demografico, attrattività dei territori, riforme fiscali, abbattimenti dei tempi della giustizia, efficienza delle infrastrutture e della pubblica amministrazione; tutto ciò che dovrebbe formare oggetto di una vera visione politica ed industriale. È questo lo sforzo richiesto dagli italiani ed è quello che stiamo provando a fare con tutte le difficoltà di un momento storico che ha messo la crisi all'ordine del giorno, molto di più che in passato. Pertanto anche con questo decreto-legge ci siamo impegnati a creare le condizioni perché tutto concorra ad un contesto solido che possa custodire e creare lavoro: questo è il fine del decreto anticipi. Un esame che non a caso si intreccia con quello della manovra. Registriamo comunque, in taluni casi, una proficua convergenza maggioranza-opposizione e da ciò derivano alcune buone norme, quali ad esempio il rinnovo del *bonus* psicologo. La Commissione bilancio del Senato ha stabilito infatti un contributo nell'importo massimo di 1.500 euro per persona, per un limite complessivo che pertanto sale da 5 a 10 milioni. È prevista poi la proroga di tre mesi, dal 31 dicembre 2023 al 31 marzo 2024, per il diritto allo *smart working* per i lavoratori del settore privato con figli minori di Arrivano anche gli aiuti per gli alluvionati della Toscana, per i quali slitta al 18 dicembre il versamento di tributi e contributi. Trova finalmente spazio anche la riforma del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Tale Fondo è uno strumento di politica economica e industriale fondamentale, che facilita l'erogazione di oltre 250 miliardi di finanziamenti. Non c'è credito senza garanzie. Il termine del *temporary framework* sugli aiuti di Stato del prossimo 31 dicembre ha reso necessario intervenire per la stabilità finanziaria e semplificazione delle piccole e medie imprese.

Insomma, il Fondo rappresenta uno strumento essenziale per favorire l'accesso al credito in una fase in cui, con l'incremento dei tassi, si intravede una stretta creditizia per le aziende più fragili. Grazie a questa norma, nel corso del 2024 potremmo quindi garantire nuovi finanziamenti per 55 miliardi di euro, mantenendo un importo massimo di 5 milioni e significative percentuali di copertura. Si introducono anche condizioni ottimali per le microimprese, con garanzia all'80 per cento per per operazioni fino a 80.000 euro tramite i confidi. Il Fondo viene esteso anche al terzo settore e, pur mantenendo il *focus* sulle piccole e medie imprese, potrà garantire anche quelle con meno di 500 dipendenti. Una riforma importante e significativa, che riconosce il valore delle piccole e medie imprese come asse portante del nostro sistema produttivo e per la quale dobbiamo ringraziare tantissimo il sottosegretario Freni e il sottosegretario Massimo Bitonci per un lavoro che è durato tanti mesi. Esprimo ancora grande soddisfazione per l'approvazione dell'emendamento a mia prima firma sull'esenzione IVA per le prestazioni di chirurgia estetica volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute o a tutelare, mantenere o ristabilire la salute anche psicofisica, ma a condizione che le finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica. L'esenzione IVA sulla chirurgia estetica curativa dimostra l'attenzione della Lega per un tema importante: la tutela del paziente che a seguito di una malattia o per altre circostanze necessita di un intervento chirurgico al fine di guarire anche dal punto di vista psicofisico, una norma di buonsenso che auspichiamo possa aiutare numerose persone. Penso in questo momento alle tante ragazzine e donne sfregiate anche in viso perché vittime di aggressione. In vista della manovra, dunque, il Governo sta cercando di dare da subito un segnale chiaro, mostrando che non si tratta di generici buoni propositi per far tornare i numeri, ma che dietro c'è una volontà, anzi un disegno, anche perché non intendiamo ristatalizzare l'economia. Nel passato, analoghe promesse si sono sprecate, quasi sempre alla stregua di meri adempimenti formali, pressoché privi di conseguenze pratiche. Oggi però i mercati hanno smesso di essere così scettici e credo che questo voglia dire qualcosa. Stiamo provando ogni giorno a fare di tutto per dimostrare di avere il pieno controllo della situazione e per mostrare che le parole non sono utilizzate alla leggera. L'aumento dell'occupazione, gli indici di borsa, lo *spread* ci confermano confermano che siamo sulla strada giusta, nonostante le tante difficoltà. La politica economica viene spesso rappresentata come un pendolo tra crescita e stabilità. La funzione principale di questo decreto e poi della manovra è garantire quella stabilità senza la quale, come senza la fiducia degli investitori,

il provvedimento che portiamo oggi in Aula attiene al decreto n. 145 del 18 ottobre 2023. In questo decreto ci sono misure urgenti in materia economica, in materia fiscale e soprattutto in favore degli enti territoriali e a tutela del lavoro e di esigenze indifferibili. Il decreto si compone di ventiquattro articoli. Nella prima parte del provvedimento si tratta il tema dell'indicizzazione delle pensioni, il tema del recupero da parte dell'INPS delle prestazioni pensionistiche indebite per i dipendenti a tempo indeterminato delle amministrazioni statali. Per le partite IVA è previsto che la seconda rata di acconto delle imposte sui redditi venga effettuata entro il 16 gennaio e senza interessi, oppure con una dilazione di cinque rate da gennaio a maggio per dare respiro a chi produce lavoro nella nostra Nazione. Si prevede lo stanziamento di 500 milioni di euro per il trasporto pubblico con rifinanziamento del fondo per il sostegno del TPL e ulteriori 35 milioni per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale. L'articolo 11, importantissimo, istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca in materia di alloggi e residenze per gli studenti universitari. L'articolo 13 finanzia con 50 milioni di euro per il 2023, la misura di sostegno per gli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese. L'articolo 14 prevede un incremento pari a 150 milioni di euro per il 2023 per il fondo relativo ad oneri derivanti dalla revoca di eventuali concessioni. L'articolo 16 ha tre incrementi importanti in ambito sportivo: Giochi olimpici di Parigi 2024, Giochi paralimpici 2024 di Parigi e Federazione ciclistica italiana. L'articolo 17 prevede 10 milioni di euro per il Fondo nazionale di politiche sociali, un tema centrale per il nostro Governo. Con l'articolo 20 si incrementa di 50 milioni di euro il contributo aggiuntivo assegnato alle scuole dell'infanzia paritaria. L'articolo 21 istituisce, presso il Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di quasi 50 milioni destinato al finanziamento di misure urgenti legate all'accoglienza dei migranti,

Sempre questo articolo, ai commi 9 e 10, reca disposizioni correlate alla crisi ucraina, con 180 milioni per la prosecuzione sul territorio nazionale del soccorso e dell'assistenza alla popolazione,

Viene confermato un emendamento importante dei relatori sul Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, quindi viene confermato l'importo massimo garantito per ogni singola impresa, con un massimo di 5 milioni di euro. Evidenzio la novità inserita per chi affitta, per brevi periodi o per finalità turistiche, immobili o porzioni di immobili e per i titolari di strutture destinate alla locazione turistica. Essi devono cioè richiedere al Ministero del turismo, per la prima volta, un codice identificativo nazionale (CIN) che va esposto all'esterno dello stabile e che deve essere indicato ad ogni annuncio pubblicato e comunicato. Questa misura è importantissima perché è finalizzata ad assicurare la tutela della concorrenza, la trasparenza del mercato e ad agevolare la lotta all'evasione fiscale nel settore; questi, sui quali il Governo si è impegnato a costruire un percorso finalizzato alla lotta concreta all'evasione e a garantire strumenti utili al raggiungimento dell'equità. Si raddoppia il *bonus* psicologo 2024, con un contributo di 5 milioni per la psicoterapia, un segnale importante per il benessere psicologico che non dev'essere un esclusivo privilegio di pochi, ma di tutti. Per questa maggioranza l'obiettivo è diffondere la cultura della salute mentale, che va garantita a tutti. In conclusione, sono stati approvati tantissimi ordini del giorno, con tante tematiche che necessitano di risposte concrete; a mia prima firma, sul tema del trattamento pensionistico per gli ex frontalieri che lavorano nello Stato di San Marino e per i quali si chiede un trattamento di parità con gli ex lavoratori frontalieri della Svizzera e del Principato di Monaco residenti in Italia, con un'aliquota del 5 per cento. Ho amministrato Coriano di Rimini,

Signor Presidente, sottosegretario Freni, onorevoli colleghi, ci apprestiamo ad approvare un importante decreto-legge recante misure in materia di pensione, di contratti pubblici, di disposizioni fiscali in favore di enti territoriali, in materia di investimenti, di sport, di lavoro, istruzione e sicurezza. A queste misure volute dal Governo si aggiunge l'importante lavoro svolto in Commissione bilancio, con l'incremento di risorse che danno risposte concrete alle attese dei cittadini. Proprio per questo importante lavoro, vorrei fare un plauso ai nostri relatori, in particolare al nostro capogruppo Claudio Borghi, perché hanno saputo ben interpretare nei lavori della Commissione tutte le richieste che vanno a toccare direttamente la vita di milioni di italiani. Cito, ad esempio, uno per tutti, semplice ma importante, l'emendamento sull'agricoltura di montagna, al fine di assicurare la sopravvivenza delle coltivazioni importanti per l'economia e il paesaggio dei territori montani, scongiurandone l'abbandono. Vorrei citare le risorse per disabili, IVA, *bonus* psicologo, proroga dell'acconto per le imposte, proroga dello *smart working* e quant'altro. Vorrei inoltre porre l'accento in particolare su un emendamento a cui, come volontario della protezione civile da più di dieci anni e come rappresentante del Friuli-Venezia Giulia in quest'Aula, tengo particolarmente. Si tratta dell'emendamento con il quale si chiarisce una volta per tutte la normativa sui volontari e coordinatori delle squadre di protezione civile per evitare che questi vengano equiparati, rispettivamente, a dipendenti o a datori di lavoro con le relative responsabilità, anche penali. La vicenda che tocca tristemente la comunità di Preone, in provincia di Udine, e tutta la Protezione civile del Friuli-Venezia Giulia, dove il sindaco e il coordinatore del locale gruppo di volontari sono stati sanzionati, con conseguenze anche penali, in seguito a un tragico incidente, aveva portato comprensibilmente tutti i volontari a bloccare le attività in segno di protesta. Ora, con questo tempestivo atto, si vuole rimettere tutti gli operatori di Protezione civile in condizioni di lavorare con maggiore serenità. Non era accettabile che chi svolge, a titolo gratuito, un'attività fondamentale per le nostre comunità dovesse sottostare a responsabilità penali e amministrative, come se fossero lavoratori subordinati o datori di lavoro. Voglio sottolineare come questo Governo, grazie alla cooperazione di tutte le forze di maggioranza, sia riuscito a dare una risposta tempestiva, assicurando una prospettiva a uomini e a donne, che, in condizioni di maltempo, di incendi e di altre calamità naturali, rischiano anche la loro vita per la nostra sicurezza e la nostra incolumità. Bene, allora, il lavoro di squadra tra Governo e Parlamento. Ancora una volta l'Esecutivo di centrodestra ha risposto in maniera puntuale, dimostrando attenzione ad una categoria, a un orgoglio nazionale ed europeo come la Protezione civile, fondamentale per le nostre comunità. Resta - signor Sottosegretario, lo segnalo a lei - da dirimere ancora una questione, relativa alle medesime responsabilità in capo ai sindaci nella loro funzione in ambito di protezione civile. Per questo motivo ho presentato un ordine del giorno che chiede al Governo di valutare queste ulteriori posizioni.

dica il contrario e cerchi ogni giorno di farci litigare. Ebbene, non ci riuscirete. Questo Governo sta dimostrando concretezza, competenza e capacità. Questo Governo rappresenta gli italiani e cerca di creare le condizioni per famiglie, imprese, partite IVA, lavoratori per poter far ripartire il nostro Paese, specialmente in un momento e in una situazione particolarmente complessi anche a livello internazionale. internazionale. Sottolineo che molto è stato fatto, ma molto ancora resta da fare. A testa bassa, a schiena dritta, lavorando sodo, vogliamo portare a casa tutti gli impegni che ci siamo presi, per noi che - amici dell'opposizione, una volta per tutte mettetevi il cuore in pace - governeremo per cinque anni,

i colleghi che in Commissione bilancio, anche nella fase delle proposte emendative a questo disegno di legge, hanno lavorato in modo proficuo e costruttivo, al fine di consegnarci oggi un testo efficace e completo, che racchiude misure volte alla riduzione della pressione fiscale, andando incontro alle esigenze delle famiglie, soprattutto di quelle più numerose, e del sistema imprenditoriale. Mi voglio soffermare su alcune misure che incidono in maniera significativa sulla quotidianità e sulla vita reale delle persone, come quelle volte alla riduzione delle aliquote da accisa sui carburanti e sui prodotti energetici, e sulle risorse destinate ai *bonus* trasporti e al rifinanziamento delle piccole e medie imprese, con la nuova legge Sabatini. Voglio anche ricordare, soprattutto ai colleghi dell'opposizione, che sicuramente non godono di ottima memoria, che il Governo Meloni, con i provvedimenti approvati e quelli che sono ancora *in itinere*, si è sempre posto un solo obiettivo - un obiettivo preminente per noi - che è quello della tutela dei cittadini e soprattutto delle fasce più deboli, quelle che voi dell'opposizione avete sempre fatto finta di salvaguardare e che, invece, nei dieci anni in cui avete governato, in maniera colpevole e intenzionale, avete dimenticato, anche quando avreste potuto risolvere i loro problemi. Siete in grado solo di inventare false battaglie ideologiche senza costruire nulla per il bene della collettività e senza, soprattutto, progettare un'idea programmatica e vincente che guardi al futuro della Nazione, perché non avete una visione politica e strategica.

che interviene sul meccanismo di rideterminazione delle aliquote d'accisa sui carburanti mediante decreto ministeriale in corrispondenza di un maggiore gettito d'IVA. La norma in esame modifica i presupposti di emanazione del decreto ministeriale di riduzione delle accise, allo scopo di condizionarlo all'aumento del greggio sulla media del mese precedente rispetto al valore di riferimento indicato nell'ultimo DEF, e non più dei due mesi precedenti. precedenti. Così come viene disciplinato con questo provvedimento, qualora si verifichi un aumento del prezzo internazionale del petrolio greggio rispetto al valore di riferimento di tale prodotto indicato nell'ultimo DEF, possono essere disposte delle riduzioni dell'aliquota di accisa attraverso l'adozione di un decreto del MEF con il Mase. Non so se vi siete accorti che i prezzi dei carburanti sono tornati ai livelli più bassi sostenibili. Ecco perché le vostre reiterate polemiche dai banchi dell'opposizione sull'incoerenza di Fratelli d'Italia sull'argomento sono palesemente demagogiche. Un'altra misura contenuta nel provvedimento in esame che mira a rafforzare e migliorare i servizi per i cittadini riguarda gli interventi sul TPL, che prevedono il rifinanziamento del fondo per il trasporto pubblico locale già istituito dal decreto rilancio, incrementandolo di 500 milioni di euro.

Sempre in tema di trasporto pubblico locale, si incrementa di 35 milioni di euro il fondo per il buono da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale e per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Tale misura si pone la finalità di agevolare i cittadini che percepiscono un reddito medio basso. quindi di un pacchetto di misure volte a incrementare e ottimizzare la circolazione dei cittadini, migliorando la mobilità territoriale. Per noi questo significa avere una visione strategica. Un altro tema affrontato nel disegno di legge riguarda le micro, piccole e medie imprese italiane per numero, fatturato e impiego di forza lavoro. Si parla del 95 per cento. Le MPMI rappresentano una struttura portante dell'intero sistema produttivo nazionale; conoscerne le caratteristiche e incentivarne la potenzialità vuol dire sapere interpretare la realtà economica di una Nazione e rilanciare gli investimenti in maniera programmatica vuol dire salvaguardare l'economia anche in tema occupazionale. È per questo che grazie alla nuova legge Sabatini si danno nuove risorse al settore imprenditoriale. Il rifinanziamento è rivolto a tutte le micro, piccole e medie imprese al fine di ottenere un significativo beneficio fiscale per gli investimenti in beni strumentali funzionali alle attività di impresa. Per noi lo Stato e il Governo hanno il dovere di supportare e incentivare le attività imprenditoriali del territorio e credere in chi, con sacrificio e dedizione, genera lavoro ricchezza e sostiene con le proprie attività, così come accade per le nostre realtà aziendali, il sistema imprenditoriale ed economico dell'Italia. Gli imprenditori vanno tutelati e aiutati. Dobbiamo uscire dalla logica tipica della sinistra che considera chi fa impresa un nemico dello Stato. Ora elencherò alcuni punti degni di nota sempre di questo provvedimento, come previsione per i titolari di partita IVA del versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi entro il 16 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento senza interessi, dilazionando il pagamento in cinque rate. poi istituiti un nuovo contributo di solidarietà per le imprese energivore e un fondo finalizzato a sostenere gli studenti universitari fuori sede, aumentando la disponibilità di alloggi e posti letto. Si è aumentato il contributo statale alle scuole dell'infanzia paritarie e si è raddoppiato il fondo per il *bonus* psicologo, con lo stanziamento di 5 milioni

l'Italia sta ripartendo: lo stiamo dimostrando con i fatti, portando a casa risultati concreti e mettendo in pratica politiche di rilancio per il sistema economico e occupazionale, in un momento storico e sociale certamente non favorevole. Continueremo a lavorare andremo avanti così, ascoltando le tante esigenze che ci giungono dal territorio per dare all'Italia le risposte che aspetta da tempo. I Governi degli *slogan* sono finiti, come pure quelli tecnici: noi rappresentiamo il Governo che vuole rimettere in moto l'economia del Paese, ma cerchiamo di farlo in maniera consapevole e razionale, pensando al futuro e assumendoci la responsabilità di consegnare ai nostri giovani un'Italia migliore e più forte. *(Applausi)*. PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Magni.

Penso ad esempio al fatto che vi sciacquate la bocca con la questione di favorire, giustamente, l'imprenditoria privata, anche femminile e giovanile.

i lavoratori che rimangono senza posto di lavoro bisognerà trovare il modo di dare loro un sussidio, ma non producono reddito. Questo è il punto: non producono reddito

Francamente devo dire che siamo di fronte a un messaggio molto chiaro, da questo punto di vista. La voglio fare breve, perché

su questa manovra, nonostante - e finisco - il lavoro che abbiamo svolto in Commissione, con grande disponibilità. Certo, dal punto di vista del metodo, abbiamo lavorato

Signor Presidente, quello che ci accingiamo ad approvare oggi è un provvedimento importante e condiviso, con misure concrete in materia di adeguamento delle pensioni al costo della vita, di rinnovo dei contratti pubblici e di disposizioni fiscali. Forza Italia ha impresso la sua impronta e il suo tratto distintivo. Siamo fieri di questo, ovviamente, e siamo fieri di aver dimostrato, ancora una volta, che per noi l'unico punto di riferimento sono gli italiani, la loro salute e il loro benessere. Pur condividendo tutto l'impianto del provvedimento, abbiamo condotto delle battaglie che consideravamo sacrosante e che il Governo ha fatto proprie. Penso *in primis* alla salute. Il Covid ha avuto effetti devastanti su tutti noi, colpendo in particolar modo le nuove generazioni, i nostri ragazzi, privati della libertà, della socializzazione, di una vita normale, della scuola come momento di istruzione, ma anche di integrazione. Le ripercussioni psicologiche derivate da tutto questo non le abbiamo sottovalutate e non le abbiamo ignorate. La cura della mente, il sostegno, l'aiuto sono essenziali e salvano tante volte la vita; ma non tutti si possono permettere cure e sostegni adeguati. È per questo che già nella scorsa legge di bilancio, grazie alla spinta propositiva di Forza Italia, il Governo aveva introdotto il *bonus* psicologo, dando l'opportunità di curarsi a chi non ne aveva i mezzi: un fondo di 5 milioni per il 2023, che recentemente è stato sbloccato, e 8 milioni dal 2024. Forza Italia si è battuta in queste settimane per aumentare il finanziamento, facendo così crescere la platea dei beneficiati. Abbiamo quindi presentato un emendamento per triplicare il fondo per il 2023, facendolo passare a 15 milioni, e quintuplicare quello del 2024, portandolo a 40 milioni. Il Governo ha fatto sua la nostra battaglia e ci è venuto incontro con un primo importante passo, approvando la riformulazione di un nostro emendamento per portare a 10 milioni i fondi per il 2023. È una vittoria? Sì, certamente. Dobbiamo accontentarci? Ovviamente no, perché siamo convinti della disponibilità futura dell'Esecutivo a trovare la strada che porti ad aumentare il fondo anche per il 2024. Essere a fianco degli italiani significa proprio questo: conoscere le difficoltà che affrontano e trovare soluzioni reali, concrete, non facendoli mai sentire soli, perché noi non ammainiamo mai le nostre bandiere; ci battiamo in un dialogo continuo e costruttivo con i nostri alleati e facciamo in modo che diventino anche le loro. Come nel caso dell'aumento della cedolare secca dal 21 al 26 per cento per gli affitti brevi, abbiamo ottenuto dei correttivi che non penalizzino quelle famiglie che non fanno delle locazioni brevi la loro vita professionale. Come? Facendo sì che l'aliquota resti al 21 per cento per chi affitta fino a trenta giorni la prima casa *(Applausi)* e salga al 26 per cento solo per chi affitta ulteriori abitazioni. Non solo: in questo decreto anticipi abbiamo anche ottenuto l'introduzione del CIN (codice identificativo nazionale) per gli affitti turistici in chiave anti-evasione per contrastare ovviamente il sommerso. Tutto questo per dire che sono battaglie sacrosante, che Forza Italia ha vinto con lo spirito di collaborazione e il dialogo costante, certamente, ma anche per sottolineare plasticamente che c'è una grande differenza fra la propaganda e il realismo. Propaganda significa raccontare ai cittadini quello che vorrebbero sentirsi dire; sbandierare ricette miracolose; illuderli anche che, con uno schiocco di dita, le soluzioni siano dietro l'angolo: in sostanza, promettere ciò che sappiamo già non sarà mantenuto. Realismo, invece, significa parlare chiaro; essere onesti; avere la diligenza del buon padre di famiglia che non solo agisce con senso di responsabilità, ma lo fa senza nascondere nulla, mostrando a tutti la realtà dei fatti, spiegando che bisogna fare i conti con il bilancio familiare, eppure, garantendo che una volta coperte tutte le spese, risparmiando, si potrà realizzare qualche obiettivo per fornire alla comunità quell'aiuto in più che dimostra attenzione e cura da parte dello Stato. È quello che fa il Governo ed è quello che ha fatto Forza Italia. Il decreto anticipi marcia in questa direzione: ha lasciato uno spazio di manovra ai partiti che compongono la maggioranza per incidere su quei temi che ritengono importanti per il benessere dei cittadini. Sappiamo che la legge di bilancio, a causa della voragine nei conti pubblici lasciata da un uso distorto del superbonus (20 miliardi all'anno di buco da coprire), a causa di norme figlie dell'incompetenza e della superficialità, ha un cammino già segnato. Il Governo, giustamente, lavora per tutelare le famiglie più in difficoltà, per aumentare le pensioni, per arginare la crisi economica, ma anche per far partire quel percorso di crescita e sviluppo necessario all'Italia per guardare con più ottimismo al futuro. Il futuro che abbiamo davanti è finalmente più luminoso. I dati di crescita macroeconomica sono positivi, oltre la media europea, e finalmente l'Italia ha iniziato a correre, a crescere e a rialzare la testa. Andiamo avanti con realismo e onestà, perché gli italiani si aspettano questo da noi e lo meritano.

Se vogliamo rivolgerci al Paese con onestà, non parliamo di buchi di bilancio dovuti al superbonus, perché in nessun documento pubblico c'è un buco di bilancio relativo al superbonus. Lo ha detto la Ragioneria generale dello Stato. Lo dice il Documento di economia e finanza e lo dice - anzi, non lo dice - la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza. Questo buco sta quindi solo nella comprensione dei fatti e dei numeri da parte di alcuni membri della maggioranza.

a mia prima firma, che è stato accolto insieme a quello di altri colleghi, sulla proroga dello *smart working* nel settore privato per i genitori di figli minori di quattordici anni e per i cosiddetti soggetti fragili. Siamo Siamo soddisfattissimi di questa proroga, anche se un po' al risparmio: avevamo infatti chiesto il 30 giugno, ma ci è stato concesso il 31 marzo 2024. Non possiamo certo dirci completamente soddisfatti, perché in questa proroga lasciamo fuori completamente tutti i lavoratori del comparto pubblico, che sono così sempre figli di serie B, invece che essere la punta di diamante di quello che dovrebbe essere il nostro Stato. Parliamo dei lavoratori che ci aiutano a svolgere quotidianamente le funzioni che dobbiamo mettere in campo e per offrire servizi ai cittadini. sicuramente lo farebbero meglio se, invece di essere implicitamente additati come fannulloni, venissero aiutati nello svolgimento del loro lavoro, anche da remoto, quando questo è consentito rispetto alle mansioni da svolgere. Speriamo che nei prossimi provvedimenti ci sia l'ulteriore l'ulteriore proroga anche per loro, per non mettere in campo disuguaglianze nel nostro Paese. Quanto al *bonus* psicologo, ovviamente siamo contenti che siano stati aggiunti 5 milioni ai fondi a disposizione per il 2023. Ci sarebbe piaciuto che il decreto-legge grazie al quale si potranno spendere questi soldi fosse stato varato per tempo e non solo alla fine dell'anno, e che la maggioranza avesse ascoltato i suggerimenti che avevamo dato anche nella scorsa legge di bilancio, quando avevamo evidenziato che, così come l'avevano modificato, il *bonus* psicologo avrebbe creato dei problemi; che le risorse messe a disposizione erano insufficienti; soprattutto, che cambiare tutto rispetto all'impianto precedente (che aveva già un suo decreto attuativo), avrebbe posto dei rallentamenti nella messa in campo delle risorse per i cittadini che ne avevano bisogno. È facile essere Cassandre quando si conoscono le cose, e infatti il decreto attuativo è arrivato tardissimo e le risorse non bastavano, tanto che avete dovuto aggiungerne delle altre. Speriamo che, durante i lavori della legge di bilancio, vi rendiate conto che anche le somme a disposizione per i prossimi anni non sono sufficienti; che la salute la salute mentale è un grave problema; e che, oltre al *bonus*, servono interventi strutturali. Anche al riguardo, le proposte da parte nostra sono già sul piatto per andare in questa direzione, come il sostegno psicologico nelle scuole e nell'università e lo psicologo delle cure primarie primarie che deve affiancare il medico di medicina generale. Penso che ormai abbiamo capito tutti quanto sia importante anche guardare al benessere psicologico e alla salute mentale per avere dei cittadini

Per fortuna l'emendamento di Fratelli d'Italia che consentiva ai condannati di svolgere incarichi pubblici nei Comuni e nelle amministrazioni locali l'avete ritirato.

innanzitutto ringraziare il sottosegretario Freni, il Presidente della 5a Commissione, i relatori e i membri della Commissione bilancio per il lavoro svolto sul decreto anticipi. Tengo a iniziare esprimendo soddisfazione per l'approvazione dell'emendamento a mia prima firma, che prevede una semplificazione per l'accesso alle agevolazioni fiscali per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli e orticoli, in allevamento, nella silvicoltura, nella piscicoltura e nella florovivaistica; consentendo, in caso di lavori agricoli effettuati su terreni condotti in affitto o in comodato, contraddistinti da particelle fondiarie di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati, site in Comuni montani ricompresi nell'elenco delle zone svantaggiate di montagna, nonché nei Comuni prealpini, pedemontani, della pianura non irrigua, che le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà attestante l'esclusiva e piena disponibilità del terreno possano essere rese e presentate anche dal solo esercente affittuario comodatario e non necessariamente - com'era nella norma attuale - contestualmente da affittuario, comodatario e proprietario del terreno. Tale modifica permette una semplificazione non da poco per chi conosce la peculiarità della montagna. Queste particelle, infatti, spesso risultano indivise o di proprietà di persone che non vivono nelle vicinanze, ma magari all'estero, quindi inducendo un grosso impegno per reperire le firme necessarie per svolgere lo sfalcio o il pascolo. Spesso, purtroppo, quando vengono fatte le norme, non si tengono in considerazione le diverse specificità dei territori e si tende a pensare norme adatte a realtà più grandi e a cui poi i piccoli devono adattarsi, rendendo difficile continuare a curare un territorio. Di questo, infatti, stiamo parlando: non si può approvare una norma sulla Pianura padana e calarla su terreni siti a 1.000-1.500 metri. Sfalciare un prato o destinarlo al pascolo significa combattere il dissesto idrogeologico; dare un'immagine pulita e curata dell'ambiente circostante, quindi anche una cartolina turistica. Eppure, spiegare la bontà di questo emendamento è stata un'impresa titanica. Eh già, perché spesso quando si parla di montagna e delle difficoltà di viverla, chi prende le decisioni la montagna l'ha vista solo in vacanza, se non addirittura in cartolina. Ricordo, dopo l'evento Vaia, quando avevo presentato la proposta sulle procedure d'urgenza e su un fondo apposito per ripristinare il bosco che, oltre ai danni della tempesta Vaia, sta combattendo ancora e viene distrutto dal bostrico, che un esponente del Governo giallorosso mi aveva derisa dicendomi: «La Testor e i suoi alberi». Poi, però, ci si riempie la bocca di *green*, e mi rivolgo soprattutto alla parte gialla.

Rimanendo nell'ambito agricolo, un altro emendamento della Lega del collega Bergesio chiarisce che le imprese agricole titolari di reddito agrario che siano anche titolari di reddito d'impresa, interessate dal rinvio del versamento della seconda rata dell'acconto al 2024, in quanto persone fisiche, titolari di partita IVA ai fini dell'individuazione del limite ricavi-compensi nel periodo d'imposta precedente, si fa riferimento all'ammontare del volume d'affari. Inoltre, l'emendamento posticipa dal 30 giugno al 30 luglio il termine della procedura. altro emendamento a prima firma del collega Cantalamessa prevede l'esenzione IVA per le operazioni chirurgiche estetiche volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute. Un emendamento vuole invece arginare il dilagante fenomeno elusivo dell'imposta di consumo e di vendita di prodotti illeciti che attualmente caratterizza fortemente sia il mercato dei prodotti liquidi da inalazione e senza combustione, sia quello dei prodotti accessori da fumo, ovverosia filtri e cartine. Un altro emendamento introduce una deroga al principio di unicità dei piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR ordinari), consentendo a ciascuna persona fisica residente in Italia di essere titolare contemporaneamente di più PIR ordinari, limitatamente ai casi in cui questi ultimi siano costituiti

all'articolo 204 del Testo unico degli enti locali. Agli enti locali basterà dare atto dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, anziché del progetto definitivo esecutivo. L'emendamento a prima firma del presidente Garavaglia prevede un contributo di un milione di euro ai Comuni con popolazione compresa fra i 6.000 e i 7.000 abitanti che hanno registrato nel 2023 una spesa per la tutela dei minori superiore all'importo spettante a titolo di Fondo di solidarietà comunale e che hanno subito per l'anno 2023 il trattenimento di una quota IMU per per alimentare il medesimo fondo non inferiore a euro 190.000. Inoltre, un emendamento, sempre del senatore Garavaglia, prevede più garanzie per i contribuenti soggetti a verifiche fiscali, con la possibilità per il contribuente di farsi assistere e rappresentare da un professionista durante le verifiche fiscali. Un emendamento della collega Minasi prevede disposizioni urgenti per la funzionalità del MOSE, finalizzate a garantire la prosecuzione degli interventi di manutenzione. L'emendamento del presidente Marti a supporto dell'industria fonografica amplia di 800.000 euro il limite massimo che consente alle imprese di ricevere il *tax credit* realizzare maggiori investimenti in artisti e giovani artisti. Inoltre, un'altra sua proposta emendativa prevede la possibilità per le istituzioni scolastiche di attingere agli incarichi temporanei di personale amministrativo e tecnico per lo svolgimento di attività a supporto tecnico finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori. L'emendamento 17.0.35 della collega Murelli integra la composizione del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS con la presenza di un rappresentante scelto d'intesa tra le quattro associazioni

sul decreto-legge, cercando di apportare miglioramenti e di dare risposte che vanno verso le esigenze dei territori. Positivo è anche l'emendamento del Governo che tutela i volontari della Protezione civile dai rischi di incorrere in sanzioni penali

sono state già descritte dai relatori. Sicuramente va messa in luce una misura voluta dalla Lega all'articolo 4, che rinvia per l'anno 2023 il versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi

l'articolo 13 rifinanzia di 50 milioni la misura a sostegno degli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, la cosiddetta nuova Sabatini.

criticata. Innanzitutto, bisogna tener presente la situazione in cui ci siamo trovati e che ci hanno lasciato in eredità i Governi precedenti. Noi abbiamo fatto una scelta, quella di tutelare le famiglie

testo che riorganizza due emendamenti - quello del Partito Democratico e quello presentato dalla vicepresidente Licia Ronzulli, che ringrazio - il Governo in questo provvedimento ha inteso raddoppiare la dotazione del cosiddetto *bonus* psicologo. Mi concentro su questo me lo consentirà, Presidente. Una misura che mette le persone, che ne fanno richiesta e hanno i requisiti per ottenerla, in condizioni di sostenere le spese di una terapia psicologica o di un percorso di recupero, certo insufficiente, ma comunque un innesco, spesso un primo *triage* che consente una valutazione che può fare la differenza nella vita delle persone. Mi consenta, Presidente, Presidente, una breve cronistoria. Ricordo ancora Sara Reale del nostro Gruppo parlamentare che si scervellava a far di conto quando il *bonus* era ancora una aurorale proposta di legge. Tale *bonus* è nato con il Governo Draghi, dove peraltro era seduta anche la Lega Nord, come approssimazione di una risposta ad una crisi amplificata dal Covid, un'ombra sull'anima degli italiani, quella della salute mentale, in particolare, ma non solo delle generazioni più giovani, le più esposte e nude in quei mesi soffocati, impauriti e distanti. psicologo nacque proprio qui in Senato, su iniziativa della senatrice democratica Caterina Biti, che ne fece una misura condivisa da tutti i Gruppi parlamentari, spinta che tuttavia non fu sufficiente e quell'emendamento svanì in una di quelle notti interminabili e buie delle manovre di bilancio che il sottosegretario Freni conosce bene. Da quello scacco scaturì però un grido, una risposta delusa da parte di migliaia di ragazze e ragazzi che ci dissero "ma come, avete approvato *bonus* su monopattini e zanzariere e della nostra salute mentale, di come stiamo noi, di come ci sentiamo non vi interessa niente?".

20 milioni di euro, che poi furono incrementati divenendo 25. La misura fu presa d'assalto con oltre 400.000 richieste. Vista però l'esigua cifra stanziata - solo 25 milioni - soltanto un decimo dei richiedenti riuscì ad avere il sostegno. Ce ne sarebbero voluti dieci volte tanto. Cambio di Governo, esecutivo Meloni, l'anno scorso di questi tempi. Il *bonus* passa dai 25, stanziati e spesi, a soli 5 milioni previsti per il 2023 e 8 per il 2024.

Basta guardare nelle nostre case, in quelle dei nostri amici, la *malaise*. Non servono le statistiche allarmanti sui giornali. La solitudine, la depressione, l'ansia, i disturbi alimentari, l'isolamento, l'autolesionismo, i tagli sulla pelle, le tendenze suicidarie, la morte in vita, la vita come morte. Eppure, Presidente, per riuscire ad ottenere i decreti attuativi per poter semplicemente presentare le domande per quest'anno (se ci fosse un partito soltanto dei decreti attuativi, vincerebbe ogni elezione) e perché il Ministro firmasse, ci sono voluti undici mesi - la tigna, mi lasci dire, del Partito Democratico - e una nuova petizione voluta da Fedez, cui va la mia gratitudine per quanto sta facendo su questo tema con una dolorosa sincerità. Oggi, finalmente, arriviamo a 10 milioni per quest'anno, ben 15 meno dello scorso anno. Vogliamo cogliere però questo piccolo segnale positivo, questo incremento, che - dico dall'opposizione - testimonia come su alcuni temi, accaduto ieri in quest'Aula sull'oblio oncologico e qualche giorno fa, sempre qui (onore al Senato), sulla violenza contro le donne, non solo si può, ma si deve lavorare insieme. insieme. Ancora uno sforzo: dal momento che in Parlamento siamo chiamati a dare ascolto come possiamo, voce come riusciamo e risorse come dobbiamo, al Governo attraverso lei, Presidente, dico quanto segue: abbiamo la manovra di bilancio nei prossimi giorni e soli 8 milioni sul *bonus* per il 2024, a fronte dei 10 recuperati per quest'anno, ne servirebbero dieci volte tanto, facciamo in modo che almeno ci sia il segno di una crescita della dotazione rispetto al 2023. per far capire che ci credete, che ci crediamo in questa misura (che ormai non è più un *bonus*, ma un fondo salute mentale, stabile e strutturale, sottratto all'affanno dell'incertezza) e che, assieme al lavoro che si sta facendo alla Camera sullo psicologo di base, dove, anche lì, con uno sforzo *bipartisan* si è arrivati a un testo unificato in Commissione, a quello che si dovrà fare che si dovrà fare sull'ascolto nelle scuole, nelle università, nello sport e sui posti di lavoro, segna un passaggio di stagione. Da quella in cui la salute mentale, a differenza di quanto avviene in tanti Paesi, resta la pietra di scarto del nostro sistema sanitario nazionale, che va protetto e difeso come la più cara delle nostre conquiste, a una nella quale la salute mentale è salute e basta, non solo più un diritto di tutti, ma un dovere per tutti noi, a cominciare da chi sta in quest'Aula, un dovere di ascolto, voce e risorse. Per questo 8 non bastano. La ringrazio, Presidente.

convertire il decreto-legge anticipi, contenente misure urgenti in materia economica e fiscale in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. Non voglio sovrappormi all'intervento dei relatori, dell'amica Maria Nocco e dei colleghi Damiani e Claudio Borghi, ma voglio richiamare alcuni aspetti che reputo importanti e impattanti, soprattutto per i cittadini e per le imprese. quindi delle posizioni politiche, che su alcuni temi sono distanti e inconciliabili, è vero però che il lavoro che è stato fatto

un primo aspetto che mi sta a cuore, i mutui agevolati che sono stati concessi ai dipendenti bancari degli istituti di credito, perché il Governo Meloni ha posto rimedio a una stortura relativa all'applicazione delle delle norme fiscali sui *fringe benefit* resa evidente e insostenibile dai continui rialzi dei tassi decisi dalla Banca

Si tratta di 70.000 lavoratori che, come ben ha evidenziato con soddisfazione anche la con questa modifica riceveranno una sorta di seconda tredicesima, senza tassazioni: questo credo sia un risultato importante da evidenziare. Ho parlato di collaborazione politica in un clima positivo ed è con soddisfazione che richiamo anche la proroga del lavoro agile nel privato per i genitori con figli minori di quattordici anni, che attualmente era in vigore fino al 31 dicembre, ma che potrà invece essere applicata fino al 31 marzo 2024.

i fondi rispetto a quelli previsti per il 2023 mediante una riduzione corrispondente dello stanziamento del fondo speciale iscritto nell'ambito del programma dei fondi di riserva e speciali del MEF. Il contributo è stabilito nell'importo nell'importo massimo di 1.500 euro per persona, per un limite complessivo che sale pertanto da 5 a 10 milioni di euro per il 2023; il limite, a decorrere dal 2024, sarà di 8 milioni di euro annui.

terapeutici, purché certificati con apposita attestazione medica, e alla riduzione dell'imposta al 10 per cento sugli integratori alimentari. È stata fatta su questo punto della facile ironia, ma vorrei ricordare invece l'importanza della chirurgia estetica correttiva e rigenerativa all'interno dei percorsi di cura e guarigione, anche e soprattutto a livello psicologico:

poi la modifica dell'articolo 12, comma 2, della legge n. 212 del 2000, grazie a cui si conferma il diritto, in capo al contribuente, di essere e rappresentato da un professionista abilitato durante le verifiche fiscali (quello che chiamiamo il fisco amico). Ciò significa quindi non costringere i cittadini ad affrontare da soli quelle che in qualche modo sono le forche caudine

PMI, con cui si introduce la gratuità dell'accesso per le microimprese, che costituiscono oltre il 95 per cento del nostro tessuto imprenditoriale. *(Applausi)*. Questa misura contribuisce a mitigare l'incremento dei tassi di interesse, che, come ha confermato anche CNA, apre a maggiori opportunità per l'intervento dei Confidi. E ancora, sempre per le imprese, c'è la proroga del termine previsto per la presentazione dell'istanza di regolarizzazione mediante riversamento spontaneo dei crediti di ricerca e sviluppo non spettanti, che ha posto dei problemi seri in in questi ultimi tempi; invece, da adesso in poi, i soggetti che hanno già presentato la richiesta telematica di accesso alla procedura di riversamento del bonus ricerca e sviluppo e non hanno ancora effettuato il versamento dell'unica soluzione o della prima rata possono revocare integralmente la richiesta entro la scadenza del 30 giugno 2024. I soggetti che effettuano la revoca hanno quindi un mese di tempo per presentare una nuova richiesta di riversamento entro il 30 luglio. Molto importante è ancora la proroga dell'accesso al 5 per mille per le ONLUS anche in assenza dell'iscrizione al RUNTS, per tutto il 2024, e la proroga di adeguamento statutario per associazioni e società sportive dilettantistiche, un mondo - permettetemelo su cui la burocrazia ha il dovere di muoversi con l'attenzione e con il rispetto che sono dovuti, se non altro, al ruolo sociale che ricoprono. E ancora, andando in modo molto telegrafico, c'è lo stanziamento di 50 milioni per il fondo emergenza nazionale e in particolare il sostegno alle imprese esportatrici della Toscana che sono state colpite dai recenti eventi alluvionali *(Applausi)*, sotto forma di contributi a fondo perduto, attingendo alle giacenze del fondo SIMEST. C'è poi la stretta sugli affitti brevi, con l'introduzione del CIN, il codice identificativo nazionale per gli affitti turistici concesso dal Ministero del turismo, e di altri obblighi in ordine alla sicurezza. Questo non significa ammorbare un segmento redditizio, che negli ultimi anni ha giocato

ormai approcciato in forma sempre più imprenditoriale. C'è poi la riassegnazione dell'affidamento delle autostrade abruzzesi A24 e A25 a Strada dei Parchi SpA, subentrando ad ANAS, salvando migliaia di posti di lavoro e e bloccando l'aumento dei pedaggi; una situazione paradossale, che era stata creata dai precedenti Governi giallorossi. E ancora la rafforzata capacità delle amministrazioni titolari del PNRR, tra cui Palazzo Chigi, ora nella possibilità di assumere personale per incarichi di vertice presso enti e istituti nazionali. Signor Presidente, siamo di fronte a un provvedimento che è assolutamente strutturato, razionale e concreto. Convertiamo in legge delle azioni che sono coerenti e importanti e che avranno delle ripercussioni positive per gli italiani e per le imprese. Non sono solo delle frasi di circostanza e di rito, ma è la fiducia e l'apprezzamento popolare nei confronti dell'operato del Governo Meloni a parlare. Anche gli ultimi sondaggi confermano una piena fiducia in Giorgia Meloni e nelle decisioni che sono state assunte da questo Governo. A rimarcare la bontà di quanto stiamo facendo c'è il giudizio degli italiani che è l'unico - lo voglio sottolineare - di cui ci importi realmente qualcosa. Continuiamo allora a guidare con coraggio e con grande senso di responsabilità l'Italia fuori dalle sabbie mobili dell'immobilismo politico di chi ora finge di avere tutte le soluzioni quando invece non le ha avute e non le ha ora, a maggior ragione. finestra"). Dichiaro chiusa la discussione generale. Come da accordi, sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 16. La

dicembre. Resta confermata per le giornate di oggi e di domani la discussione del decreto-legge recante misure in materia economica e fiscale. La prossima settimana sarà dedicata prevalentemente ai lavori della 5a Commissione sul disegno di legge di bilancio. L'Assemblea, tuttavia, tuttavia, si riunirà martedì 12 dicembre, alle ore 16, per i seguenti argomenti: votazione a scrutinio segreto mediante schede per l'elezione di un senatore Segretario; mediante schede)* - Consegna del testo delle Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2023 2023; discussione del decreto-legge su disposizioni per gli uffici presso la Corte di cassazione in materia di *referendum*, già approvato dalla Camera dei deputati. Il giorno successivo, ovvero mercoledì 13 dicembre, alle ore 9,30, si terrà la discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 14 e15 dicembre 2023.

La Conferenza dei Capigruppo potrà essere convocata prima dell'inizio della seduta del 18 di dicembre. Comunico che, in attesa che la Commissione bilancio completi i propri lavori, sospendo la seduta fino alle ore 17,30. La seduta è sospesa.

reciproco che ci dobbiamo, non solo per il lavoro quotidiano che facciamo, ma anche per gli impegni che assumiamo

il decreto-legge anticipi, l'unico decreto-legge dell'impianto complessivo della manovra che ha avuto anche gli emendamenti della maggioranza, sia finito in una strada senza uscita; quella strada dei tentativi continui della maggioranza stessa e del Governo di modificare alcune materie sulle quali la stessa maggioranza non ha avuto né il coraggio né l'ordine da parte del Governo di intervenire nel disegno di legge di bilancio. Io penso che ci sia un limite che non si deve mai superare ed è stato superato quando il Governo, il giorno della conferenza stampa sulla legge di bilancio,

È stato fatto dicendo in maniera roboante al Paese che, siccome la maggioranza era coesa e compatta, non avrebbe presentato emendamenti. Noi vi abbiamo detto sin dal primo momento che su temi di rilevanza nazionale, a partire dalle pensioni, arrivando alla casa, agli affitti, al mercato tutelato, alle alluvioni di Toscana, Emilia Romagna e di tutte le Regioni che sono state colpite, ai temi sociali, chiedevamo semplicemente di essere ascoltati per provare a far cambiare idea alla maggioranza, che in alcuni casi, almeno nei corridoi, nelle Commissioni, quell'idea l'ha cambiata. Poi se c'è o meno il coraggio per cambiare posizione, lo vedremo quando voteremo gli emendamenti.

hanno convenuto di ritirare buona parte degli emendamenti del decreto anticipi, proprio per consentire al Governo un confronto serio su alcuni di questi temi. Il risultato è che siamo alle ore 19,10 e arrivano arrivano ora gli ultimi emendamenti, che noi contestiamo, che i nostri colleghi hanno contestato in Commissione bilancio. È inaccettabile, che il Governo abbia perso tempo su code di condoni e su pseudo rottamazioni e che non ci dia ancora risposte sulle pensioni. Oggi abbiamo scoperto che forse domani arriveranno gli emendamenti del Governo sulla legge di bilancio, che diranno che restano tutte le iniquità della riforma sulle pensioni, che forse toccano qualcosa delle fasce dai sessantasette a settant'anni. È in ballo la vita delle persone. Ci sono 730.000 lavoratori italiani che stanno aspettando una risposta da quest'Aula. Signor Presidente, quella risposta non arriverà nemmeno stasera. Allora la nostra proposta è di iniziare domani mattina, di analizzare meglio le proposte emendative arrivate per l'Aula qualche minuto fa, come potrà testimoniare il Presidente della Commissione bilancio. Avremmo comunque concluso i nostri lavori alle ore 20. Prendiamo dunque i 50 minuti per approfondire il merito delle modifiche apportate in Commissione bilancio e domani mattina riprendiamo i lavori, sperando di ritrovare la maggioranza e il Governo meno confusi di come li abbiamo trovati in questi giorni.

abbiamo esaminato in discussione generale qualche ora fa, per il quale ci accingiamo, oggi o domani, a votare gli emendamenti per l'Aula, tratta della conversione in legge di un decreto del 18 ottobre 2023. Non siamo alla terza lettura. Il decreto del 18 ottobre arriva in Aula il 6 dicembre, per la totale incapacità di Governo e maggioranza di gestire un percorso che, grazie alle forze di opposizione, è stato assolutamente ordinato. Non c'è stato un momento di ostruzionismo in Commissione bilancio, neanche un momento. dovevamo ricominciare - lo dico come esempio - alle ore 16,50 i lavori in Commissione per dare il parere sugli emendamenti. Abbiamo ricominciato alle ore 18,30 e siamo in Aula alle ore 19, perché non arrivava il parere sul testo A

come si possa pensare di arrivare in modo ordinato a discutere la legge di bilancio. Aggiungo che, nonostante i lunghi tempi di discussione in Commissione bilancio, non c'è stata la voglia di discutere di un ennesimo condono, che questo Governo e questa maggioranza stanno proponendo e che è contenuto nell'emendamento 4.0.300, del quale noi chiediamo il ritiro, per ridare dignità a quest'Aula e perché il provvedimento possa continuare in modo ordinato la sua conversione. Credo sia necessario un atto di responsabilità da parte delle forze di maggioranza che stanno sostenendo l'ennesimo condono.

richiesta avanzata dal presidente Boccia e per utilizzare questo spazio per una riflessione, che parte da una constatazione. Come è stato ricordato, questo provvedimento arriva in fondo senza attività ostruzionistica da parte delle opposizioni, senza che vi sia stato da parte nostra un atteggiamento di non cooperazione con la normale dialettica parlamentare e anche all'insegna di un dialogo che abbiamo avviato sul piano procedurale e metodologico con tutti i Gruppi e con il Governo, finalizzato a interpretare anche questo provvedimento

qualche difetto di fabbrica, diciamo così. Il primo difetto di fabbrica, politicamente tutto in capo alla maggioranza, è dato dal fatto che, con una scelta assolutamente originaria, la maggioranza ha deciso di non far presentare ai propri componenti parlamentari emendamenti alla legge di bilancio. Il risultato è che il provvedimento Il risultato è che il provvedimento oggi al nostro esame è stato infarcito di interventi, proposte ed emendamenti che i colleghi della maggioranza avrebbero avuto tranquillamente la possibilità di far transitare nella sede naturale, quella cioè della legge di bilancio. Aggiungo anche con l'arrivo all'ultimo momento, secondo un malvezzo dal quale sembra che inevitabilmente non riusciamo ad emendarci; cambiano le maggioranze, ma non cambiano i cattivi costumi degli arrivi all'ultimo momento di proposte fuori sacco, sulle quali non vi sono i pareri della ragioneria, che costringono la Commissione bilancio a delle rincorse costanti e ansiogene,

attenzione perché il calendario rischia di andare in cortocircuito esclusivamente per vostra responsabilità e non per responsabilità delle opposizioni. Oggi, signor Presidente,

sicurezza e copertura del rinnovo contrattuale del comparto sicurezza; un tema su cui noi dall'opposizione avevamo detto che bisognava intervenire e sul quale ora vogliamo vedere cosa è stato scritto. Si riscrive il tema della previdenza; si interviene sugli enti territoriali e - udite, udite - è in arrivo un pacchetto di nuove opere pubbliche che dovrebbero essere finanziate - non si capisce bene decise come, dove e da chi - e all'interno di esse l'inevitabile, immarcescibile e tradizionale Ponte sullo Stretto di Messina, che ancora una volta viene fatto oggetto di un intervento legislativo. Capite bene che, se questo è il metodo con il quale noi ci approcciamo all'interno della legge di bilancio,

che non hanno fatto ostruzionismo, ma per mera, esclusiva e piena responsabilità della maggioranza, rischia di andare in cortocircuito. A questo punto a me pare che la proposta avanzata dal presidente Boccia sia assolutamente condivisibile al fine di consentire domani un naturale e anche lineare percorso di approfondimento degli emendamenti e degli ordini del giorno per i motivi che ho detto in precedenza - motivi che fanno parte di un ragionamento complessivo con l'approvazione, nei termini che avevamo preso secondo gli impegni con il ministro Ciriani, entro la giornata di domani.

un rapporto corretto tra maggioranza e opposizioni. Non solo non abbiamo fatto ostruzionismo, ma addirittura abbiamo accettato un'impostazione tale il Governo ci aveva detto di affrontare le risposte, quindi di individuare gli emendamenti che si definivano ordinamentali e quelli onerosi. Abbiamo accettato un percorso,

in cui si interviene su materie delicate, come diceva prima il presidente Patuanelli.

però facciamo una cosa come questa: si presenta un emendamento che è un condono da una parte e, dall'altra, si interviene su una materia pensionistica o sulla questione dello sport

ma abbiamo già visto cose molto simili. Detto questo, siccome dobbiamo organizzare i lavori, credo che sia ragionevole iniziare domani, perché adesso, quando arriverà il parere scritto della Commissione bilancio i cui membri tutti ringrazio, a cominciare dal presidente Calandrini, per il lavoro che svolgono ogni giorno - dovrà essere annotato, pertanto non potremmo iniziare nei prossimi minuti e avremmo davvero poco tempo. Ritengo pertanto ragionevole iniziare domani,

Ci sono dei tempi che i Gruppi devono utilizzare, ma quelli sono i tempi assegnati; arriveremo quindi in modalità ragionevoli al voto e alle dichiarazioni di voto. Non mi pare che il Governo abbia messo la fiducia; quindi chiedere chiedere un approfondimento è assolutamente utile. Non si deve nemmeno far sì che poi il Governo si contraddica, avendo detto che non mette la fiducia, cosa che tecnicamente potrebbe fare, ma non fa, per favorire l'illustrazione degli emendamenti e delle posizioni principali, come è stato detto dai Capigruppo, però con orari e modalità che siano in linea con un lavoro normale. Se diciamo all'esterno che cominciare alle 9 è strano, non credo che la gente la prenderebbe bene; anzi, si potrebbe cominciare anche prima. Ci sono dei tempi previsti dal Regolamento. Possiamo quindi domani concludere regolarmente la discussione in maniera ordinata, senza voto di fiducia, ma con l'esame di merito, come è stato auspicato più volte.

Ho parlato troppo presto sulla comunità di intenti. C'è una metà che chiede alle 9 e una metà che chiede alle 9,30.